Signor Presidente, onorevoli senatori, riferisco oggi in Senato in qualità di Ministro della salute su una vicenda che mi coinvolge anche dal punto di vista personale, in quanto fino a tre anni fa ho operato come medico e ricercatore dell'Ospedale San Raffaele, ancorché in convenzione prima con l'università Statale e poi con l'università Milano Bicocca. Vorrei, quindi, premettere all'esposizione della vicenda così come vista dal punto di osservazione del Ministero della salute, alcune mie considerazioni personali.

e perseguire la «missione» con la massima determinazione. Don Luigi Verzé ha entrambe queste doti. Ha una *vision* straordinaria ed è poi estremamente determinato ed efficace nel perseguire gli obiettivi che si prefigge. È stato uno dei primi a riportare in Italia i cosiddetti cervelli in fuga emigrati all'estero. Anch'io sono tra questi. Ha così messo in piedi una struttura sanitaria, il San Raffaele, con uomini di prim'ordine, motivati da emulazione e al tempo stesso da spirito di corpo che hanno ottenuto a partire dagli anni Ottanta e Novanta risultati scientifici e clinici di assoluto rilievo internazionale, facendo «volare» il nome del San Raffaele in tutto il mondo. Un grande successo italiano. Affermatosi che fu l'Ospedale milanese, don Verzé si dedicò ad altre iniziative: i grandi laboratori di ricerca di base a Milano, strutture sanitarie all'estero e successivamente altre attività sempre più variegate ed eterogenee rispetto all'iniziativa originaria. Onorevoli senatori, ecco cosa ci può essere stato alla base delle attuali difficoltà finanziarie del San Raffaele: una grandissima forza realizzativa che ha creato un'opera unica nel nostro Paese, ma che a un certo punto si è trasformata in una sorta di spinta a crescere in modo autonomo e non più direttamente correlata agli obiettivi di partenza. Resta il fatto che l'Ospedale San Raffaele, con i suoi 4.000 medici, ricercatori, tecnici, infermieri e amministrativi è e resta una struttura straordinaria in cui si fa della straordinaria assistenza e ricerca clinica, una struttura che non si può neppure pensare di non difendere e mantenere come grande patrimonio nazionale. Fatte queste mie considerazioni personali, veniamo ora al punto di vista del Ministero della salute. Il San Raffaele è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico La normativa vigente definisce gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità». Le competenze del Ministero della salute sono mirate al riconoscimento di tale carattere, sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge, ed alla vigilanza, che consiste prevalentemente nella verifica triennale del mantenimento dei suddetti requisiti. Nello svolgimento di tale attività, la legge prevede che, in presenza di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata come il San Raffaele, deve essere fatta salva «l'autonomia giuridico-amministrativa» dell'istituto. Restano estranei ai compiti del Ministero la regolazione, la gestione e il controllo dei rapporti con il sistema sanitario, che rientrano tra le competenze della Regione, così come non rientrano tra i compiti del Ministero interventi di qualsiasi natura o attività di vigilanza sugli assetti societari, sulle attività extrasanitarie e su quelle estere: attività che appaiono oggi all'origine del forte indebitamento della fondazione. Avendo appreso dagli organi di stampa della difficile situazione finanziaria della fondazione, delle scelte gestionali del suo consiglio di amministrazione e successivamente della tragica, e per me assai dolorosa, scomparsa dell'ex vicepresidente, Mario Cal, il Ministero ha richiesto all'Istituto e alla Regione Lombardia un dettagliato rapporto in ordine alle difficoltà finanziarie e agli interventi sulla *governance* dell'Istituto. Infatti, la stabilità finanziaria è una delle condizioni per garantire il corretto svolgimento dell'attività di ricerca, di assistenza e di didattica, nonché il corretto uso dei finanziamenti per la ricerca, erogati a favore degli IRCCS, che non possono certamente essere utilizzati per altri fini che non siano quelli di ricerca. In questo contesto problematico, va comunque sottolineata l'assoluta eccellenza scientifica e sanitaria del San Raffaele e anche l'equilibrio finanziario ad oggi delle mere attività sanitaria e di ricerca. I costi dei 1.083 posti letto dell'ospedale, per circa 57.000 ricoveri l'anno, più l'attività ambulatoriale e quella clinico-universitaria, sono coperti dai contributi della Regione Lombardia e delle altre Regioni (considerato che quasi un terzo dei ricoverati non sono cittadini lombardi), che nel 2010 hanno erogato al San Raffaele complessivamente 390 milioni di euro. Anche l'attività di ricerca è in equilibrio finanziario: nel 2010 i finanziamenti hanno superato i 54 milioni di euro, provenienti da varie fonti pubbliche e private, italiane e internazionali, come il Ministero della salute, la fondazione Telethon, la fondazione Cariplo, l'European research council e il National istitute of health statunitense. Questa è la migliore conferma dell'eccellenza della ricerca del San Raffaele, che "produce" 700-800 pubblicazioni scientifiche l'anno e ha avuto nel 2009 un *impact factor* (l'indice che misura l'attività di ricerca) pari a 3.923,83, il più alto fra i 43 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico italiani e tra i più alti in Europa fra tutti i centri di ricerca. Del resto, come ho già segnalato, le origini dell'indebitamento appaiono estranee ai settori della ricerca e dell'assistenza sanitaria. Oggi si tratta di fare luce su questi aspetti e, nell'interesse dell'Ospedale, non posso che esortare tutti i responsabili del San Raffaele, a cominciare da don Luigi Verzé, a cui mi legano sentimenti di profondo affetto e gratitudine, a collaborare pienamente con i nuovi amministratori. Ai nuovi consiglieri di amministrazione, espressione di realtà sanitarie di eccellenza e di istituzioni finanziarie e imprenditoriali di area cattolica, e ai loro consulenti spetta il compito di arrivare a un quadro chiaro della situazione contabile e la responsabilità di elaborare un efficace piano di ristrutturazione nei termini concessi dall'autorità giudiziaria, al fine di proseguire l'alta missione dell'Istituto. Lasciano ben sperare le recenti dichiarazioni di disponibilità di esponenti di istituzioni bancarie creditrici del San Raffaele, che sono essenziali per continuare a garantire la liquidità per l'attività corrente in queste delicate settimane. Il Governo continuerà dunque a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda, pronto a operare, nell'ambito delle proprie competenze, per favorire la messa in sicurezza delle attività sanitarie e di ricerca del San Raffaele, da ritenersi un patrimonio irrinunciabile per il nostro Paese.

signor Ministro, anzitutto la ringrazio per essere venuto qui a riferire su una vicenda che rischia di privare l'Italia di uno dei maggiori centri sanitari di eccellenza. Un'eccellenza riconosciuta in tutta Europa. Un'istituzione le cui benemerenze in capo scientifico, al di là di qualunque valutazione di altro tipo, non possono essere negate. In questi giorni abbiamo letto di tutto sui giornali: piantagioni brasiliane, palazzi e ospedali nei Paesi dell'Europa orientale, aerei ed elicotteri intestati a società della Nuova Zelanda. Centinaia di milioni di investimenti improbabili che hanno messo sul lastrico un colosso sanitario. Ma, a dire il vero, forse si poteva intuire che qualcosa non andava già guardando semplicemente all'Italia. Forse, ha suggerito qualcuno, ancor più semplicemente ai dintorni di Milano. Pensiamo alla Costa Smeralda, ad esempio: niente ospedali, niente opere di bene. Più prosaicamente un hotel a quattro stelle, riservato a una clientela d'*elite*, di proprietà della Fondazione Monte Tabor. La Fondazione ha dirottato milioni di euro dalle attività sanitarie a quelle alberghiere che peraltro, a quanto emerge, non avrebbero neppure dato utili. Tutto sommato una piccola cosa, almeno se confrontata con il miliardo e più di debiti che grava sul San Raffaele, ma che riesce a dare un'idea di come, con l'andar del tempo, una miriade di investimenti con scopi non proprio filantropici e di progetti megalomani ha minato alle fondamenta una grande opera a favore della collettività, con il contorno anche di evidenti conflitti di interessi. Ingenti finanziamenti sono stati in parte assorbiti da altre iniziative che nulla avevano a che fare con il bene comune, come, ad esempio, la colossale cupola con l'arcangelo sulla sommità, che troneggia sull'edificio principale del San Raffaele, costata oltre 60 milioni di euro. Ma anche speculazioni immobiliari come quella a Cologno Monzese dove una società del San Raffaele ha restaurato una villa storica immersa in un parco dove ha anche costruito decine di appartamenti. Anche qui adesso tutto è fermo: invenduti gli appartamenti, fin qui proposti a prezzi giudicati fuori mercato, e la società oberata dai debiti e posta precipitosamente in vendita. Tutto ciò impiegando gran parte degli oltre 400 milioni versati ogni anno dalla Regione Lombardia per i rimborsi dei medicinali e dei ricoveri in convenzione: cioè con i soldi versati dai cittadini contribuenti. Per un po' il peso di questa strategia folle è stato fatto ricadere sui fornitori. E così il debito verso le aziende che riforniscono il San Raffaele, dalle aziende farmaceutiche a quelle informatiche, è esploso fino a superare i 500 milioni. Ciò che è più grave, e che va sottolineato con forza perché è il vero problema di questa vicenda, è che il dissesto della Fondazione Monte Tabor sta provocando un danno innanzitutto alla collettività che non vedrà realizzate quelle che invece erano le opere di utilità sociale. A Cologno Monzese, ad esempio, dovevano essere costruiti e consegnati al Comune un ristorante e un *auditorium*. I lavori sono attualmente fermi ed è probabile che così resteranno. Ad Olbia è stato costruito un nuovo ospedale che è costato oltre 200 milioni di euro. Una struttura certamente utile in una Regione con una situazione sanitaria non certo felice come la Sardegna, finita di costruire pochi mesi fa e che sembra però destinata a restare ferma fino a quando non si chiarirà il destino dell'intero gruppo sanitario San Raffaele. In tutta questa vicenda, signor Ministro, chi ha pagato finora, e rischia di pagare anche in futuro, sono i cittadini: siano essi i contribuenti della Regione Lombardia e dell'Italia tutta che rischiano, dopo aver pagato per anni milioni di euro di rimborsi, di perdere i servizi e le prestazioni di una grande struttura ospedaliera e i vantaggi di un'importante struttura di ricerca, siano essi gli imprenditori e i dipendenti delle aziende fornitrici che rischiano di non vedere onorati i propri crediti, oltre che i ben 3.700 dipendenti dello stesso San Raffaele che rischiano il proprio posto di lavoro. A questo punto, signor Ministro, è necessario porsi quantomeno un interrogativo: la Regione Lombardia, che in questi anni ha versato con puntualità assoluta (come dovrebbe essere, del resto) i rimborsi dei medicinali e dei ricoveri in convenzione, e il Ministro della sanità hanno vigilato affinché questo denaro pubblico, cioè dei cittadini, fosse effettivamente impiegato a favore dei cittadini stessi? E quante strutture o gruppi sanitari privati convenzionati sono oggi nella stessa situazione del San Raffaele? Accertare come sia stato possibile creare una simile voragine finanziaria ed individuare le eventuali responsabilità è un compito che spetta alla magistratura, ma alla politica e alle istituzioni spetta il compito di assicurare la necessaria trasparenza nelle procedure affinché tali situazioni non abbiano più a ripetersi. *(Applausi

mai negata alla sua persona, che non ho ben capito le cause del disastro di questa struttura sanitaria e scientifica, che è una delle eccellenze italiane.

della comunità nazionale, soprattutto per alcune malattie, che qui erano e sono egregiamente curate. Pertanto, preciso subito che l'obiettivo non è quello di strumentalizzare questa vicenda per alcun fine,

di debiti sia dovuta ad altre attività, che non sono quelle di ordine sanitario. Va effettuato assolutamente un controllo e posto riparo a questo disastro, che

Signor Ministro, dobbiamo salvaguardare assolutamente quest'istituto. Questa è la mia opinione, e credo di interpretare anche quella di diverse componenti del Gruppo Misto. Dobbiamo salvarlo, come una delle più grandi eccellenze della sanità italiana, e inserirlo nel progetto, di cui tante volte abbiamo discusso, di una rete di eccellenze in Italia, che dovrebbero appartenere anche alle altre Regioni. Ma di questo magari

lavora e fa ricerca, di tutte le persone che sono state curate - come la sottoscritta - o che sono tuttora in cura. Ma per poter fare questo - mi spiace, signor Ministro - quello che lei oggi ci ha riferito non è sufficiente, quanto dobbiamo occuparci di chi non ha esercitato la sua responsabilità di controllo, ma anche di chi ha tradito le finalità sanitarie e di ricerca proprie di una struttura come questa. I problemi del San Raffaele investono tre aspetti: la magistratura, l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario e i livelli sanitari e di ricerca. Quanto alla magistratura è grave, gravissimo, che si sia arrivati a questo, che si sia accumulato un deficit ingente e si siano effettuati investimenti che esulano dalla finalità dell'ente stesso. La Fondazione Monte Tabor non avrebbe dovuto investire risorse in operazioni che non corrispondono al fine iniziale: farsi carico della salute della persona umana senza conseguire fini di

a lei e al suo Ministero nel suo insieme, come ha fatto a non controllare in modo adeguato questo IRRCS e quali controlli ha fatto la Regione. Compete al Ministero della salute controllare la Regione se non effettua i controlli, visto che non solo ha accreditato, ma anche convenzionato questa struttura, e quindi utilizza soldi della fiscalità generale. Ma il San Raffaele è una fondazione, un ente non commerciale e non ha mai chiesto la qualifica di impresa sociale. Non era obbligato a presentare i bilanci in prefettura, avvalendosi della riservatezza contabile: un meccanismo che può funzionare per le piccole fondazioni, ma non per il San Raffaele. Se ci fosse stato un reale e sostanziale meccanismo di controllo, anche attraverso lo strumento della *due diligence,* ovvero dell'attività necessaria per analizzare lo stato dell'azienda e i rischi di un eventuale fallimento, il vaso di Pandora si sarebbe aperto prima e non ci saremmo trovati in questa situazione. Il Governo non può delegare queste azioni all'iniziativa facoltativa dei privati. Le fondazioni, per chi le parla e per la forza politica che rappresenta,

Compete al Parlamento il dovere di approvare in tempi rapidi una legge sulle fondazioni e una revisione del decreto legislativo sulle imprese sociali. Serve però anche una revisione della legge istitutiva dei DRG, ma prima ancora, o mentre il Parlamento compie queste scelte, il Ministero ha l'obbligo di fare quei controlli che finora sembra siano stati effettuati in modo non sufficientemente efficace, e di controllare per quale

San Raffaele, a quella nobile e preziosa tradizione che è stata tramandata lungo i secoli: quella tradizione che deriva dal cristianesimo in campo sanitario. È sufficiente ricordare il Fatebenefratelli, il Cottolengo, le Ancelle, i Camilliani,

intervento le parole di un santo, Giuseppe Moscati, che era anche un medico: «Se la vita può essere definita un lampo nell'eterno (...), la medicina si assuma la responsabilità di una sublime missione». Se il Parlamento, il Ministero e le Regioni svolgono la loro

acqua che disseta e spada che divide il bene dal male. Qui vale proprio la pena di dividere il bene dal male. Serve quindi un'indagine dettagliata, e lo chiediamo a lei, signor Ministro, le cui risultanze puntualmente dovranno essere riferite all'interno del Parlamento.

Signor Ministro, ho apprezzato molto la sua relazione, e anche il passaggio di natura personale. Credo che la vicenda riguardi la sua storia, per cui capisco davvero il suo sentimento.

desiderato e voluto - e quella *mission* hanno avuto una spinta autonoma a crescere: in biologia è ciò che qualifica la cellula neoplastica, quella che cresce senza controlli. Questo è accaduto. Qualcuno che doveva controllare non ha controllato. Lei ha raccontato quali sono i compiti del Ministero, che conosciamo. Penso Penso che in questa vicenda non possa sussistere un atteggiamento in alcun modo notarile. Se il Ministero deve riconoscere quei caratteri che danno la scientificità alle istituzioni e deve verificare, deve anche verificare costantemente che siano integre le possibilità di assicurarle all'interno di una struttura virtuosa. Non vorrei, davvero non vorrei - e lo dico anche da persona,

Nazione e che i pazienti debbano essere tranquillizzati sul fatto che continuerà ad eccellere, perché ne ha tutte le potenzialità.

così significativa anche nel nome, per molti di noi, ci si aspetta una virtuosità particolare, e non di scoprire che alcune attività sono compatibili solo perché non si pagano i fornitori da 500 giorni.

pur avendo, come lei stesso ci ha detto, signor Ministro, una particolare attenzione proprio per la storia che in questa istituzione ha avuto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare in maniera particolare il ministro Fazio per questa informativa

Inoltre, non dimentichiamoci che il tutto é arrivato alla ribalta delle cronache in seguito ad un episodio a dir poco tragico, il suicidio del vice presidente, dottor Cal,

stiamo parlando di una struttura particolarmente importante. Non vorrei esagerare nel reputarla infatti la migliore eccellenza sanitaria nazionale e tra le più importanti

non facciamoci nemmeno lontanamente prendere dall'idea di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Le cose sono completamente diverse. Al limite, credo che questa vicenda possa aprire un ulteriore orizzonte di dibattito - e in questo caso il Parlamento è sicuramente una sede seria e competente per cercare di rivedere i criteri di gestione e di finanziamento degli istituti di ricerca a carattere scientifico rispetto alle aziende ospedaliere sanitarie che fanno capo ai sistemi sanitari regionali.

è che si possa proseguire in questa *mission* e questa *vision* di cui lei stesso, signor Ministro, ha parlato sulla scia dell'illuminato don Luigi Verzé, che si possa proseguire nel portare avanti il buon nome e la buona azione del San Raffaele nel senso

Nonostante questo, le avrei chiesto maggiore chiarezza sulla situazione e sulle prospettive del San Raffaele. Il tema vero è capire perché questo istituto abbia accumulato un debito così a quanto pare non in rapporto alle attività di istituto di carattere sanitario per le quali il San Raffaele viene pagato con denaro pubblico, ma, secondo le notizie che circolano in questi giorni, in rapporto ad altre attività che nulla avevano a che fare con questa missione. Tra l'altro, questa situazione rischia di trascinare nel baratro anche altre istituzioni prestigiose, come l'Università del San Raffaele (tre facoltà, 2.000 studenti)

allo statuto proprio in questi giorni, i componenti del consiglio di amministrazione dell'università saranno nominati da don Verzé, cosa che consentirà a quest'ultimo di controllare anche nei prossimi anni la vita dell'ospedale, dato che gli stessi docenti sono anche i primari della Ha preoccupato molto anche noi il silenzio della Regione Lombardia, che tra l'altro ha portato molte volte il metodo San Raffaele come metodo virtuoso da contrapporre al pubblico inefficiente ed inefficace e prendiamo atto del fatto che lei ha chiesto un rapporto alla Regione Lombardia. Vorrei dirlo però anche ai miei colleghi: questo non giustifica affatto la questione. Non si può dire che la responsabilità è solo degli enti che non hanno vigilato, anche se noi non assolviamo nessuno, né la Regione né il Ministero. Ma la responsabilità prima è dell'istituzione che, come qui spesso è stato ripetuto,

2006 fa obbligo a chi vuole fregiarsi di questo titolo di depositare i bilanci civilistici e consolidati alla Camera di commercio: questo avrebbe fatto sì che i bilanci del San Raffaele fossero sottoposti allo scrutinio di banche, fornitori, giornalisti, opinione pubblica, e forse qualcuno avrebbe potuto accorgersi prima della grave situazione che si andava determinando. Essendo tra l'altro l'istituto di cura e ricerca San Raffaele senza scopo di lucro, questa qualifica di impresa sociale sarebbe stata un elemento di garanzia, non solo per tutti cittadini che si curano nella sua struttura, ma anche per tutti coloro che versano il 5 per mille ogni anno in suo favore nell'ambito della loro denuncia dei redditi. Quindi, signor Ministro, chiedo, anche a nome del mio Gruppo,

di *ticket* (addirittura ci sono *ticket* previsti nel 2014, oltre a quelli già applicati che appesantiscono la spesa privata, anche di persone indigenti), di fronte a questa chiamata a sostegno di una situazione difficilissima per il Paese da parte delle persone più disagiate, io credo che non possiamo essere in nessun modo indulgenti verso chi usa il denaro pubblico per altri obiettivi che non quelli propri e per chi lo

intanto per aver risposto immediatamente alla richiesta formulata qualche giorno fa in quest'Aula dalla collega Bassoli e dal sottoscritto volta a sapere dal Ministro quali iniziative si intendessero prendere a garanzia del San Raffaele. Signor Ministro,

Nel 1982 avveniva il riconoscimento quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor. C'è un intervento concreto.

c'è un nuovo consiglio di amministrazione composto da personalità del mondo sanitario e del mondo economico di altissimo livello, quali il professor Profiti, presidente dell'ospedale Bambino Gesù,

letto, per un totale di 1.397 posti letto. Ma non è solo questo. Bisogna ricordare che questa struttura nel 2010 ha effettuato 53.000 ricoveri, oltre 8 milioni di prestazioni ambulatoriali, oltre 25.000 interventi chirurgici ed oltre 65.000 accessi al pronto soccorso. Dobbiamo trovare modi e termini affinché questa struttura, la sua professionalità, il suo valore, non solo per la Lombardia ma per l'intero sistema sanitario nazionale, siano garantiti. Noi, onorevole Ministro, la ringraziamo di questo intervento, di questo controllo. Non vogliamo porre all'indice nessuno,

una serie di interventi che andavano invece indirizzati sempre più all'istituto di ricerca e cura a carattere scientifico. Va ricordato, inoltre, che vi operano 3.292 dipendenti e 453 consulenti, che le facoltà di medicina, di chirurgia, di psicologia e di filosofia hanno 1.860 iscritti.

Non mi piace la risposta data qualche giorno fa dai magistrati al professor Flick che era andato a chiedere tempi lunghi per

che questa struttura rimanga un valore del Servizio sanitario nazionale, che possa rappresentare un faro della ricerca. Lei ha ricordato poc'anzi il rientro dei cervelli e quanti di questi operatori, di questi ricercatori operano all'interno di quella struttura. senza quella struttura tanti cervelli non sarebbero tornati, tanti operatori non sarebbero diventati il fiore del sistema sanitario nazionale e del sistema sanitario regionale.

perché anche il nome del San Raffaele era una presa di posizione storica e culturale. Ricordo che Raphael vuol dire medicina di Dio, Dio Dobbiamo verificare che il nuovo consiglio di amministrazione con l'intervento pubblico, con l'intervento della Regione, con l'attenzione del Ministero della salute sia in condizione di operare affinché si seguiti a lavorare

per garantire che si possa seguitare a lavorare nell'interesse del nostro servizio sanitario, dei ricercatori, ma anche delle 8 milioni di prestazioni offerte nel 2010 da una fondazione che deve seguitare a vivere, nell'interesse comune.

Onorevoli colleghi, come preannunciato ieri alla Conferenza dei Capigruppo e successivamente comunicato all'Assemblea, la Presidenza ha proceduto all'armonizzazione dei tempi per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2567 per complessive nove ore

ieri durante la lettura del calendario di questa settimana e della prossima, ma ci saremmo aspettati, come accade solitamente, che si concludesse la fase preliminare che stiamo svolgendo, e cioè l'illustrazione e poi la votazione delle questioni pregiudiziali e della questione sospensiva. Non si capisce perché il procedimento

manca poco, credo solo tre interventi, a concludere la fase preliminare. Peraltro, sottolineo che è noto il potere del Presidente cosiddetto di armonizzazione, cioè di regolazione dell'andamento dei lavori in modo tale da poter arrivare a una conclusione entro l'arco temporale più o meno indicato, ma altra cosa è il provvedimento che lei ci ha letto adesso. Il provvedimento che lei ci ha appena comunicato non è un'armonizzazione, signor Presidente, è un contingentamento dei tempi, che costituisce materia riservata alla Conferenza dei Capigruppo. Quindi, le chiedo espressamente di convocare la Conferenza dei Capigruppo al fine di vagliare la possibilità di contingentare i tempi. Si tratta di un provvedimento, signor Presidente, che non ha nessuna urgenza, lo abbiamo sottolineato più volte, e non si capisce perché,

modificare o revocare questa decisione, oppure di convocare la Conferenza dei Capigruppo, perché lei ci ha indicato il contingentamento dei tempi, che è cosa diversa dall'armonizzazione dei tempi. intervengo per associarmi alla richiesta del collega Legnini. Presidente, lei oggi all'apertura della seduta, subito dopo l'informativa del ministro Fazio, ci ha sostanzialmente comunicato il contingentamento di questo provvedimento. Non si tratta di armonizzazione: a nostro avviso - mi trovo assolutamente d'accordo con quello che ha detto il senatore Legnini - siamo in presenza di un contingentamento, che spetta, come le assolutamente noto, alla Conferenza dei Capigruppo. Anche a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori le chiedo la revoca di questa decisione della Presidenza, formalmente le chiedo di convocare la Conferenza dei Capigruppo perché non riteniamo assolutamente possibile che questo provvedimento

del senatore Legnini e dell'Italia dei Valori e per chiederle di convocare subito la Conferenza dei Capigruppo.

voglio ricordare che ieri alla Conferenza dei Capigruppo il nostro Gruppo ha chiesto l'armonizzazione dei tempi e, quindi, i colleghi che hanno partecipato

ha tutta l'autorità e le prerogative per assumere le sue decisioni, ma la questione ieri era stata da noi correttamente posta alla Conferenza dei Capigruppo, come mi

come la calendarizzazione approvata all'unanimità nella precedente settimana, non è un fatto sorprendente: sono cose di cui abbiamo già discusso e che abbiamo anticipato e che la Presidenza si era riservata di comunicare all'Aula in base all'andamento della discussione. Dico questo per ristabilire la verità dei fatti, per chi c'era.

il processo penale italiano, e al Gruppo del Partito Democratico sono stati assegnati un'ora e venti minuti di tempo per i suoi interventi. Lei mi dica come si possa chiamare armonizzazione questa decisione della Presidenza! Noi le chiediamo di poter discutere

debba illustrare tutti gli argomenti a sostegno della tesi che definisce questo provvedimento probabilmente il peggiore, rispetto al processo penale, dell'intera legislatura; Presidente, non è in nessun modo accettabile che, burocraticamente, ci venga tagliato il tempo per discutere. Noi siamo minoranza in questo Parlamento, e sappiamo quali sono le regole dei rapporti tra maggioranza e minoranza, ma vogliamo il tempo per discutere, e lo vogliamo in proporzione all'importanza e alla delicatezza degli argomenti che si trattano. La Presidenza del Senato deve rispettare la minoranza, e lo deve fare perché questa è la regola principale principale di ogni democrazia. Se voi non rispettate i nostri diritti, questa discussione rischia in modo consistente di degenerare. Prego quindi la Presidenza di assumere con responsabilità una una decisione seria sulla distribuzione del tempo per la discussione del provvedimento che stiamo esaminando e la ringrazio molto, signor Presidente, perché sono certo che lei avrà apprezzato apprezzato gli argomenti che le abbiamo esposto e che prenderà decisioni conseguenti. La prego di non far proseguire,

del fatto che l'Aula deve poter lavorare serenamente, e questa decisione non dà serenità all'Aula. La ringrazio. vorrei mantenere i toni su un buon livello. Presidente Gasparri, armonizzazione non significa contingentamento: anzi, armonizzazione significa cercare di trovare una sintesi tra le diverse richieste. Abbiamo dimostrato anche in passato un in passato un comportamento che è stato sempre lineare, il più possibile propositivo, ma abbiamo chiesto di avere i tempi giusti per poter parlare,

se su argomenti di questo genere, che già hanno un *vulnus* di origine, proviamo

non colmabile delle opinioni, è un conto; se invece la maggioranza e la Presidenza del Senato intendono, se non esasperare, quantomeno non venire incontro alle nostre richieste, ognuno se ne assume la responsabilità, anche quella di approvare un provvedimento "fetecchia" alla vigilia della pausa estiva.

simuli, sotto forma di armonizzazione, un vero e proprio contingentamento dei tempi. Sarebbe stato più logico, nonché più utile ai fini di una discussione serena, considerato che abbiamo un decreto-legge in scadenza, consentire al Senato di esaminarlo prioritariamente, senza costringere l'Assemblea a tempi estremamente ristretti nella discussione di questo provvedimento, che comunque - come i colleghi della maggioranza sanno - non sarà esaminato dalla Camera

logica, salvo il riconoscimento implicito di una debolezza politica interna alla maggioranza, che sa bene che la Lega non voterà mai questo provvedimento provvedimento dopo l'approvazione del decreto rimpatri. In questa logica è comprensibile quello che i colleghi della maggioranza stanno facendo: non è condivisibile, non è corretto e non è giusto, ma lo posso capire. Ma se questo non c'è, e, come affermano loro stessi, la maggioranza è compatta, non c'è il problema di una trattativa tra la Lega e il PdL sui temi che riguardano la sicurezza e la giustizia, non vedo la ragione per la quale non non possiamo utilizzare il tempo necessario per esaminare a fondo la conversione del decreto-legge che riguarda i temi della sicurezza e posticipare l'esame

Colleghi, capisco tutte le argomentazioni di questo mondo, ma mi sembra che ieri il Presidente del Senato comunicato che avrebbe armonizzato i tempi della discussione in relazione al modo in cui si sarebbe svolta e al numero degli interventi.

apertura rispetto alle ragioni Il Presidente del Senato in quell'occasione ha fatto chiaramente riferimento ad una valutazione che avrebbe effettuato in concreto quando l'argomento fosse venuto in discussione, con ciò dimostrando che voleva riservare all'attenzione dei Gruppi più tempo

in maniera chiara ed evidente che avrebbe armonizzato i tempi in relazione al numero degli interventi, la mia decisione non può che essere conseguente*.(Commenti dai

Io sono sempre comprensivo nei confronti dei ragionamenti di tutti, ma voi vi renderete conto che il nostro compito è quello di rispettare il Regolamento, e io ritengo che su questi temi il Regolamento sia ben chiaro, sia con riferimento all'esercizio del contingentamento ai sensi dell'articolo 55, comma 5, sia con riferimento al potere di armonizzare i tempi, che, presidente Belisario, è esplicitamente previsto qualora non scatti il contingentamento. Ritengo che il Presidente del Senato sia stato attento alle ragioni delle opposizioni: se, infatti, si fosse deciso per il contingentamento,

e consentito che nella discussione, rispetto ad una decisione della Presidenza, comunque si ascoltassero più voci dello stesso Gruppo. Per un richiamo al Regolamento adesso ascolto lei, presidente Legnini, ma capirà che la Presidenza è obbligata a prendere le sue decisioni. lei poco fa ha detto che, come è noto, è tenuto a far rispettare il Regolamento. La comunicazione che ci ha fatto, e che ora ha confermato,

quando il Presidente compie una valutazione dell'economia complessiva dell'andamento dei lavori, e così via, allora indica ai Gruppi la necessità di attenersi ad una scadenza, ad una data, ad un giorno, esercitando un potere che sta dentro e non oltre il calendario deciso

e la Lega Nord si assuma la responsabilità di far esaminare prima quest'obbrobrio di provvedimento del processo lungo e poi il decreto-legge a firma del ministro Maroni sui rimpatri: da tre anni ci stanno facendo «'na capa tanta» su questi rimpatri e allontanamenti, e oggi sono

Presidente Legnini, le confermo quanto ho già dichiarato. Le aggiungo che già ieri il Presidente del Senato, durante i lavori d'Aula, ha annunciato testualmente che: «Per quanto riguarda il disegno di legge in materia di giudizio abbreviato

contiene un'espressione che lei ha omesso, e cioè che "per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina" e poi Quindi, siccome si tratta di un potere della Presidenza che è già stato esercitato, lei capisce, presidente Legnini, che non posso assolutamente, rispetto ad una prerogativa esercitata dalla Presidenza, venire meno. In ossequio alla interpretazione sistematica da sempre seguita in questa Assemblea, il potere di organizzazione previsto dall'articolo 84 del nostro Regolamento è prerogativa della Presidenza, non soggetta a discussione non soggetta a discussione né a richieste di votazioni. *(Commenti dal Gruppo PD.)* Ciò tra l'altro si evince dal fatto che tale potere può essere esercitato se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione

ha detto ciò che lei ha letto, ma ha detto anche un'altra cosa molto importante, e cioè che avrebbe adottato provvedimenti atti ad armonizzare e ristabilire il clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Questo lo abbiamo annullato. Ciò che mi interessa di più, dal punto di vista procedurale, è un altro elemento:

PdL).* Signor Presidente, lei ci ha appena detto che non può rimettere in discussione una determinazione del Presidente del Senato, che aveva già comunicato la sua volontà di procedere all'armonizzazione

Non era scontato che il calendario sarebbe stato confermato dall'Aula. Noi abbiamo immaginato di poter convincere i colleghi a cambiare il calendario retrocedendo questo provvedimento rispetto al decreto sui rimpatri. Oggi che ciò non è avvenuto, riteniamo di non accedere all'idea di armonizzazione; ma se deve esserci, che sia contingentamento in Conferenza dei Capigruppo, assumendo in pieno questa responsabilità. Mai si è dato il via libera ad un'armonizzazione dei tempi rispetto al fatto che la nostra richiesta era quello di

deciso a maggioranza - ovviamente le opposizioni erano contrarie - il contingentamento. La Presidenza, per dare più spazio agli argomenti dell'opposizione,

l'ultima volta che ho controllato il nome delle nostre istituzioni ancora ho trovato scritto "Parlamento", quanto meno dal punto di vista formale, per cui parlare è l'unica cosa che c'è rimasta. Lei ha interpretato una decisione per la quale ci vengono contingentati i tempi su qualcosa che non è né necessario né tantomeno urgente,

il Parlamento è fatto per parlare e per dire ciò che non va , nel merito e nel metodo, va cercando di mantenere, allo stesso tempo, anche il rispetto per se stessi. Qui il rispetto per se stessi è sceso a nota a piè pagina dei nostri lavori quotidiani proprio per il modo con cui si concede, mi sia consentito,

Qualunque decisione non può annullare ciò che gli uffici hanno già ufficializzato.

significa tornare indietro rispetto a quello che è già ufficiale. Significa che non possiamo più parlare nemmeno sugli emendamenti! Significa che vi vergognate del provvedimento e volete soffocare la libertà di

non posso parlare neanche un minuto e mezzo. Allora, un principio di ragionevolezza nel contingentamento, che salvaguardi i diritti individuali dei senatori deve essere garantito dalla Presidenza. È irragionevole la proposta che sta facendo la Presidenza: é in violazione dei miei diritti personali come rappresentante degli elettori lombardi.

relativamente agli articoli 93 e 55, ricordando in quale momento della discussione su questo disegno di legge Noi stiamo ancora esaminando le questioni pregiudiziali e le richieste di sospensiva, per cui non abbiamo ancora dato inizio alla discussione generale. generale. Siccome non è stato ancora posto il problema dell'iscrizione di tutti i nostri senatori e la partecipazione alla discussione generale, credo che non sia ancora possibile in questo momento contingentare i tempi. Siamo in una fase del tutto preliminare rispetto a quella che è regolamentata dall'articolo 55

si sarà in grado di valutare se vi sarà una discussione generale e quali dovranno essere i tempi per la stessa, eventualmente da contingentare o da armonizzare. Aggiungo poi un argomento specifico a queste mie osservazioni.

che l'Aula sia messa in grado di valutare la legittimità costituzionale anche di questo nuovo emendamento aggiuntivo per riproporre la questione della stessa legittimità costituzionale. Solo all'esito di questa, saremo in grado di votare sui profili preliminari costituzionali e sulla questione sospensiva, per poi cominciare la discussione generale. Per questo motivo, credo sia quanto mai opportuna una riunione della Conferenza dei Capigruppo per valutare questo emendamento aggiuntivo, i nuovi profili di legittimità costituzionale e poi i tempi successivi per la discussione generale.

intendevo rendermi garante del corretto e pacifico andamento dei lavori anche su temi conflittuali e non condivisi, e questo intendo fare. Io intendo mantenere l'impegno assunto in Conferenza dei Capigruppo all'unanimità, che è quello di andare in vacanza dopo aver approvato i testi individuati nel nostro calendario approvato all'unanimità e gli argomenti deliberati, che sono quelli a voi noti.

intervenendo sul contingentamento dei tempi, se necessario. Poiché però voglio fugare qualunque ipotesi di critica o di preoccupazione da parte dell'opposizione per cui io intenda strozzare il dibattito su un tema del genere, anche se ieri avevo anticipato che sarei intervenuto sull'armonizzazione,

assumo responsabilmente la scelta, ora per allora, di adottare in prosieguo qualunque provvedimento di contingentamento finalizzato a rispettare l'esecuzione del calendario approvato all'unanimità, che prevede l'approvazione del decreto-legge sull'immigrazione, l'approvazione di questo testo, l'approvazione di un altro disegno di legge ordinario, che voi conoscete e che ho citato, ed eventualmente l'approvazione delle ratifiche - questo, entro la giornata di giovedì della prossima settimana

dei provvedimenti, alla luce delle vostre manifestazioni di dissenso, proprio per fugare qualunque strumentalizzazione, seppure in buona fede, da parte di qualunque esponente dell'opposizione, revoco il provvedimento di armonizzazione, al fine di consentire all'Aula di continuare il dibattito che si era incardinato su questo provvedimento, di terminare l'illustrazione delle questioni pregiudiziali, votarle, accettarle o respingerle, e continuare iniziando la discussione generale. riservo ovviamente ulteriori valutazioni, determinazioni e decisioni nel prosieguo dei lavori per garantire un principio, che entro giovedì della prossima settimana questo calendario che voi conoscete venga totalmente ripulito - scusate l'espressione - nell'esame di questi testi di legge.

andamento dei lavori. Convocheremo naturalmente altre Conferenze dei Capigruppo, ma ribadisco che resta fermo l'impegno di questa Presidenza, da un lato, di essere garante dei diritti dell'opposizione e, dall'altro lato, di essere garante del rispetto del calendario, approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo che vede l'approvazione di questi disegni di legge

l'orientamento dell'opposizione di impedire l'approvazione di questo provvedimento. PRESIDENTE. Lei può essere contrario. Impedire mi sembrerebbe un'espressione un po' forte,

c'è qualcosa nel dibattito che non funziona. Il Presidente deve presiedere l'Aula, non deve battibeccare con i senatori che intervengono. Lei mi ha dato la parola: mi lasci parlare. Lei ha parlato di una sua intenzione di far approvare questo, questo e quest'altro provvedimento, ed io le ho risposto che noi cercheremo di impedirlo perché lei non doveva dire che voleva far approvare il provvedimento. Lei deve regolamentare i lavori, non far approvare i provvedimenti. *(Applausi

un provvedimento che reca e ha ad oggetto la inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, ma nel corso del suo esame e, segnatamente, a seguito dell'approvazione di una serie di emendamenti, anzi di un emendamento approvato dalla maggioranza, questo provvedimento è cambiato totalmente, per cui dal punto di vista formale e sostanziale è un'altra cosa. Le chiedo allora di volere esaminare, alla luce delle questioni pregiudiziali che abbiamo posto, anche questo profilo di natura regolamentare che attiene all'articolo 97 del nostro Regolamento, perché è evidente che un conto è essere chiamati qui a votare un provvedimento che riguarda un argomento

Grazie, signor Presidente. Sarò brevissimo, per consentire al Presidente di partecipare alla cerimonia funebre. Voglio ricordare che avevamo deciso all'unanimità un calendario. Questo fatto non lo dovete scordare.

di un provvedimento (lo ha detto con un tono che non era quello di uno che annuncia solo un voto contrario), prendiamo atto della decisione che il Presidente ha motivato in maniera molto responsabile nella volontà di non turbare il clima costruttivo dell'Aula su un calendario che è stato approvato all'unanimità. Voi avete il diritto di opporvi, noi abbiamo il diritto di sollecitare la discussione e la votazione e di auspicare l'approvazione di un provvedimento che, tra l'altro, traspone letteralmente i principi dell'articolo 111 della Costituzione, e che quindi difendiamo anche nel merito. *(Applausi

Questo benedetto calendario approvato all'unanimità è stato inserito nello *speech* con un numero e un titolo completamente diverso dal contenuto del provvedimento. di fronte alla provocazione di qualcuno che mi ha detto che dovevo ricordarmi a memoria il numero (perché siamo stati provocati proprio nella Conferenza dei Capigruppo), ho risposto

Grazie,

Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni rispetto alla nostra proposta di non procedere

appaia contradditorio, difforme, direi forse anche irragionevole rispetto all'impostazione della politica del Governo sulla giustizia, esplicitata anche in sede formale dal Ministro della giustizia in più di un'occasione. politica che, per la verità, per quanto attiene o atteneva alla diagnosi, ci ha visti anche in alcune circostanze concordi, magari non sulle terapie ma sull'analisi. Cos'è stato ricordato in questi tre anni, signor sottosegretario Caliendo? Qual era il punto di vista della maggioranza? In questo Paese i processi sono troppo lenti, le procedure sono troppo lunghe e abbiamo la necessità di riportare i tempi della giustizia entro

di ridurre i tempi dei processi, di sospendere i processi, di interrompere i processi e di fissare per legge un termine entro il quale il processo, se non arriva una sentenza di primo grado, di appello o di Cassazione,

tutta un'azione che avrebbe dovuto avere come obiettivo l'evitare che il nostro Paese fosse condannato, così com'è accaduto, dalla Corte di giustizia Grazie, del processo una delle condizioni che contraddistinguono un ordinamento come rispettoso dei diritti stessi delle persone e dei cittadini. mi pare che siamo ad un'inversione della rotta, ad un repentino cambiamento. Si potrebbe quasi parlare di "contrordine compagni": il processo non deve più essere breve, ma lungo. Si potrebbe dire che il processo deve essere sufficientemente lungo per essere in alcuni casi tempestivamente breve. Quello che voi ci proponete è non solo in contrasto con l'articolo 101 della Costituzione, ma è contraddittorio rispetto ad una linea seguita fino ad oggi. Il processo deve essere breve o deve essere,

cosa vi sia di rispettoso nell'interesse generale della ragionevole durata del processo in questo provvedimento.

le modifiche agli articoli 190 e 495 del codice producono un'estensione del processo che non è nemmeno calcolabile. Possiamo dire che è indeterminata perché il numero dei testimoni che potrebbero essere sentiti non è ragionevolmente prevedibile. sembra non tener conto non solo dell'interesse dell'imputato che dovrebbe vedersi riconosciuto in tempi ragionevoli l'accertamento intorno alle sue responsabilità, responsabilità, ma neanche degli interessi delle altre parti nel processo, ovvero della parte offesa ovvero, se vi è, della costituzione di una parte civile, perché, di fronte a un processo che si dilata nel tempo, credo che l'interesse ad avere giustizia in tempi celeri e ragionevoli non è più una certezza acquisibile. L'effetto è ancora più grave se si considera la circostanza che, in base al comma 5 dell'articolo 1, la nuova disciplina si applica anche ai processi in corso per i quali, alla data di entrata di in vigore della legge, non sia stata disposta la chiusura del dibattimento di primo grado. Non è una norma procedurale all'interno di una revisione organica del processo, ma addirittura è una novella che va ad intervenire dentro i processi che sono in una fase processuale aperta e che sono, quindi, all'esame e in discussione. È altrettanto difficile comprendere come possa conciliarsi

in materia di acquisizione a fini probatori delle sentenze passate in giudicato, secondo cui le prove che hanno portato ad assumere circostanze e fatti come sufficientemente dimostrati e che sono dentro un provvedimento passato in giudicato non possono più essere utilizzate, secondo un normale

nella direzione di raggiungere nei tempi più brevi possibili l'accertamento della verità e della responsabilità: irragionevole modifica, per non dire uno snaturamento, del regime di ammissibilità delle prove nel processo penale, collocata in un provvedimento che, come si è detto più volte, in origine aveva lo scopo, anche interessante e per certi versi condivisibile, di regolamentare il rito abbreviato per quanto riguarda i reati punibili con l'ergastolo. All'interno di questo provvedimento si è invece inserita una norma che nulla

sul regime dell'ammissibilità della prova che, evidentemente, fino ad oggi si ritiene non abbia ben funzionato e non abbia garantito una normale ed efficiente acquisizione di elementi probatori. Per queste

consentito dal Regolamento adeguato a dare una risposta ad una violazione straordinaria e palese del nostro Regolamento. Per la verità,

ritenendo improponibile la materia oggi in esame perché in netta

Non si tratta solo di un cavillo formale, cioè la risposta a una tecnica di produzione normativa

Infatti, la norma dell'articolo 97 tutela la sostanza della regolarità del procedimento legislativo parlamentare. Non può e non deve accadere che giunga in Commissione o in Aula un provvedimento con un contenuto definito al quale sia apposto successivamente, con una contorsione del suo contenuto, un provvedimento che non è vicino o appena lontano dall'oggetto, bensì tutt'altra cosa. Tutt'altra cosa, infatti, è la materia della inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo rispetto delle prove durante il processo di primo grado. Non vi è alcun nesso, nessuna connessione, neppure una lontana interferenza.

su un argomento diverso da quello sul quale avevamo concentrato la nostra attenzione. A causa di questa violazione, si è generato un provvedimento i cui effetti, ancora una volta, non siamo in condizioni di determinare, questa improvvisa modifica del contenuto fa mancare alla discussione l'analisi sugli effetti. Quanti sono i procedimenti in primo grado che non si sono conclusi e che possono avvalersi di questa norma? Quant'è il tempo di prolungamento di quei procedimenti? Come si incrocia questo allungamento con i tempi attuali della prescrizione? In sostanza, accelera o rallenta i tempi per giungere alla conclusione del procedimento?

i processi sono troppo lunghi e si arriva ad una decisione quando la stessa ha perso i suoi effetti nella maggior parte dei casi e, nell'altra ipotesi, per più del 15 per cento dei procedimenti penali incardinati non si arriva ad un esito definitivo perché intervengono i tempi della prescrizione, sia ordinaria che processuale. Questo provvedimento genera una riduzione di questi fenomeni, di entrambi, o una loro accentuazione? Non ci sono elementi, neppure nelle relazioni di chi ha avanzato la proposta, che ci confortino sul primo versante: anzi, tutti gli argomenti militano a sostenere la nostra tesi in base alla quale avremo una lievitazione delle percentuali di processi prescritti. E il processo prescritto è la peggiore soluzione, il peggior epilogo dell'attività giudiziaria in campo penale, perché nega l'aspirazione alla giustizia. Tenete conto che non sempre è lo Stato che si contrappone all'imputato: nella gran parte dei processi è un cittadino che vuole vedere ristorato

tenacemente orientato a questa relazione, lo Stato che ce l'ha con gli imputati eccellenti, introduciamo una norma che nega la giustizia anche nella relazione tra cittadino e cittadino. Quindi, per coprire la prima ipotesi o la prima categoria noi neghiamo giustizia giusta ai cittadini nelle loro relazioni.

corpo l'altra ragione, cioè la violazione dell'articolo 111 della Costituzione. Il Costituente ha posto un limite all'attività normativa,

introduce spazi e finestre che sono dilatori rispetto alla conclusione del procedimento stesso, smarrendo quindi l'effetto che è garantito. Insistiamo quindi con molta forza perché il provvedimento non passi all'esame

la copertina porta un titolo mentre il contenuto è un altro. Se il sistema editoriale volesse emulare il sistema normativo,

Bisogna trarre le conseguenze da un atteggiamento e da un orientamento che non appartiene alla maggioranza o alla minoranza, ma che dimostra che l'opinione pubblica è stanca di un Parlamento che tratta

Colleghi, così non si può continuare. Vi prego di allontanarvi dall'Aula o di ascoltare in silenzio. Prego, Grazie, signor Presidente.

come funziona la disciplina dell'Assemblea e come, in relazione alle necessità di funzionamento di un'Assemblea o di un contesto pubblico di un contesto pubblico di questo genere, chi presiede possa e debba avere i poteri per garantire il funzionamento. E questo mi sembra interessante notarlo, perché il provvedimento di cui oggi discutiamo e in ordine ai cui gravi profili di illegittimità costituzionale

dobbiamo essere estremamente chiari: con l'approvazione di questo disegno di legge, il processo penale italiano viene tecnicamente cancellato dall'orizzonte costituzionale e istituzionale. E la prego di considerare, signor Presidente, che io tendo a pensare le parole che adopero, quindi se faccio un'affermazione di questo genere è perché ben presenti le conseguenze che, letteralmente, dal giorno dopo l'approvazione di una normativa siffatta verrebbero a determinarsi nelle aule di giustizia italiane. Fra poco cercherò di illustrarvi tali conseguenze con per rendere comprensibile anche ai non addetti ai lavori come il vizio di legittimità costituzionale rischi di inverarsi, anzi certamente si invererà in una disfunzione totale dell'apparato penale italiano se questa legge dovesse essere approvata. Ma, come ho detto, questa esemplificazione la offrirò fra poco. Adesso voglio soffermarmi brevemente sulle ragioni testuali che ci inducono ad affermare... *(Brusìo).*

che ci inducono a ritenere in termini di certezza la sussistenza del vizio denunciato con la questione pregiudiziale. Discutiamo, anzi discuteremo, ove la questione pregiudiziale non fosse accolta e quindi si passasse all'esame del provvedimento, fra le altre cose della nuova formulazione dell'articolo 190 del codice di procedura penale. Molto interessante e significativo ai nostri fini è quel passaggio della nuova norma la quale recita l'imputato ha diritto all'acquisizione "di ogni altro mezzo di prova a suo favore" mentre le altre parti "hanno le medesime facoltà in quanto applicabili». Il giudice, in base a questa norma, verrà obbligato ad ammettere - a pena di nullità, sia chiaro

Questo significa che, se fosse approvata la norma cui ora mi sto riferendo, il giudice sarebbe obbligato, a pena di nullità, ad ammettere prove manifestamente superflue o irrilevanti. Ci insegnano, infatti, i professori e gli studiosi di teoria del diritto e dell'interpretazione che uno dei criteri criteri fondamentali per la corretta interpretazione delle norme è quello dell'analisi della volontà del legislatore e una lettura comparativa dei testi di legge, quando un testo sia modificativo di un testo precedente. Quindi, se nella norma precedente si la facoltà per il giudice di non ammettere le prove manifestamente superflue o irrilevanti e questo riferimento viene eliminato, il significato dell'operazione normativa è esattamente questo: voi volete che il giudice sia obbligato ad ammettere le prove manifestamente superflue o irrilevanti. Veniamo rapidamente ora a un primo punto di contatto, e quindi a una prima riflessione, in ordine alla questione articolata di legittimità costituzionale che stiamo proponendo. Esiste una possibilità di tenere nello stesso argomento, esiste cioè un profilo di compatibilità concettuale e costituzionale, fra il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 111 della Costituzione e il principio dell'obbligo di irrilevanza previsto dall'articolo 190 così come vorreste modificarlo? Naturalmente la domanda è retorica: non esiste nessuna possibilità di tenere nello stesso orizzonte di coerenza concettuale e argomentativa queste due nozioni, che sono antitetiche. È impossibile, rispettando un principio costituzionale che impone la ragionevole durata del processo, quindi una nozione superiore di ragionevolezza, coordinare l'obbligo dell'irrilevanza.

pratica, in concreto cosa accadrebbe dopodomani - un dopodomani ipotetico che io spero non venga mai -, nel momento in cui questa normativa dovesse essere applicata. caso ci occorre una lettura delle norme del codice di procedura penale e del codice penale in materia di oggetto della prova e di come si raggiunge la prova su certe questioni fondamentali. Perdonate dunque la pedanteria, ma vi leggo l'articolo 187 del codice di procedura penale, che così recita: «Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza». La La determinazione della pena e della misura di sicurezza è oggetto di prova, e quindi rientra, a pieno titolo, nella fattispecie dell'articolo 190, quello attuale e quello che sarebbe modificato, quindi rileva in questa prospettiva la individuazione dei criteri sui quali il diritto alla prova si esercita, e ancora di più si eserciterà in futuro, attraverso i quali considerare la gravità del reato ai fini della valutazione e quantificazione della pena. Questo è l'articolo 133 del codice penale, che voglio leggervi perché sia ben chiaro quello che potrebbe ipoteticamente succedere Recita l'articolo 133 del codice penale: «Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione, 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo». Allora, uno potrebbe chiedersi, non essendo addetto ai lavori: perché il senatore Carofiglio ci legge questo articolo? Perché ogni singola... *(Richiami del Presidente).* La ringrazio, Signora Presidente. Arrivo rapidissimamente alla conclusione. Ogni singolo profilo di cui all'articolo 133 del codice penale è soggetto a prova e potrà essere provato utilizzando materiale probatorio irrilevante o manifestamente superfluo, con una sostanziale ablazione della potestà punitiva dello Stato. Per questo motivo sussiste una grave contraddittorietà di questo testo con l'articolo 111 della Costituzione, e quindi chiedo

Alla Camera il 17 febbraio 2011 fu approvato un disegno di legge che era molto chiaro ed esplicito: disciplinare l'impossibilità di ricorrere al rito abbreviato nei procedimenti relativi ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. una buona base di partenza, la possibilità di confrontarsi con un testo per far in modo che per alcuni reati gravi punibili con l'ergastolo non potesse essere ammesso il rito abbreviato. Al Senato abbiamo guardato questo testo con interesse. Il Gruppo del Partito Democratico presente in Commissione giustizia era pronto a migliorarlo, ad emendarlo. In noi prevalevano le preoccupazioni che il testo potesse recare dei danni alla lotta alla mafia e anche ad altri reati particolarmente gravi. gravi. In modo particolare, volevamo prestare attenzione al ruolo dei collaboratori di giustizia e volevamo che fossero esclusi per incentivare il loro contributo, facendo riferimento non solo ai reati di mafia ma anche a quelli di terrorismo e ad altri particolarmente gravi. Poi é stato introdotto il virus della legge *ad personam*, un disgraziato e potente virus, e la legge ha subito una mutazione. ha subito una mutazione. che ha distrutto il vecchio testo, facendo nascere una nuova realtà normativa che ancora una volta mira a raggiungere il risultato che tutti conosciamo: togliere dai guai processuali il Presidente del Consiglio. Insomma, un testo di legge costruito per migliorare, almeno nelle intenzioni della Lega,

che ancora una volta mortifica le culture giuridiche del nostro Paese e gli approcci diversi alla politica giudiziaria e al sistema di sicurezza, comprime

la legge *ad personam* deve caratterizzare tutti i testi di legge che fanno capolino, sia alla Camera che al Senato.

e si faceva notare che anche i moderati, gli elettori del centrodestra, hanno detto no a un utilizzo del Parlamento per inserire leggi *ad personam* Anche i vostri elettori hanno compreso che questo meccanismo é devastante e negativo e lede i diritti fondamentali dei nostri cittadini ad avere giustizia.

mortifica, anche all'interno della stessa maggioranza, chi vuole offrire un contributo sincero e libero da strumentalizzazioni al miglioramento del processo penale nel nostro Paese. Ecco perché la Lega perde consenso. Ecco perché sarà sempre più difficile, all'interno del centrodestra, comporre questa contraddizione. Ecco perché è necessario rimuovere la causa principale, il ruolo del Presidente del Consiglio alla guida di una maggioranza che non può più sopportare il peso di un'impostazione sulla giustizia che ancora una volta le impone di volare basso, che ancora una volta la costringe a svolgere una funzione molto perdente, ma anche molto misera e disonorevole all'interno delle Aule del Parlamento. Lo stesso testo, signora Presidente in questa mutazione, ha dovuto travolgere il Regolamento del Senato,

assecondare questa impostazione, si macchia di una gravissima responsabilità, perché il buon andamento dei nostri lavori e la correttezza della gestione del rapporto tra maggioranza e opposizione richiedono una vigile attenzione alle norme regolamentari e una

È evidente la violazione anche delle nostre norme costituzionali. Di volta in volta si utilizza il processo corto

condanna o di assoluzione che sia. L'obiettivo finale è sempre quello che tutti conosciamo, la prescrizione, la cancellazione cioè del processo, dell'esigenza di avere una giustizia avere una giustizia in tempi ragionevoli, in grado di valorizzare al massimo la formazione della prova in dibattimento e nel contraddittorio delle parti. Signora Presidente, non mancano approcci culturali, non manca nelle democrazie avanzate la necessità di porre in relazione chi gestisce il potere con la giustizia, e in tutte le democrazie, le grandi democrazie, questo problema si è posto. Si è posto il problema dello *status* del principe o del sovrano quando lo scettro è passato al popolo, al popolo sovrano, appunto. Tutte le democrazie hanno sperimentato, valutato, realizzato un meccanismo di bilanciamento dei poteri, soprattutto quando hanno dovuto rafforzare gli Esecutivi e consentire così alla politica di avere un ruolo decidente,

Qui in Italia, nell'Italietta, si è fatto in modo del tutto diverso. Quando si è chiesto più potere per gli Esecutivi, parallelamente si sono chiesti più privilegi e più impunità, ma abbiamo avuto un'altra deriva, che la maggioranza oggi palesemente manifesta, che si è stati anche disponibili a sacrificare le necessità di rafforzare gli Esecutivi pur di avere un rapporto con il potere in grado di coniugarsi con più privilegi e più impunità. Ecco perché, signora Presidente, nel lo si è voluto e in questa legislatura - e anche oggi nell'incontro del Presidente del Senato con i giornalisti si richiamava la necessità di avere alle spalle una legislatura costituente - si è fallito; ecco perché, signora Presidente, noi diciamo chiaramente che c'è una violazione palese dell'articolo 111 della nostra Costituzione.

che il nostro Paese ha pagato a caro prezzo, e che è nata dopo le stragi di Capaci (Falcone) e via D'Amelio (Borsellino). Ecco perché,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, parlo a favore delle questioni pregiudiziali e sospensiva sollevate in quest'Aula a proposito di un provvedimento la cui natura non esito a definire ignobile. Le illustrazioni delle questioni pregiudiziali e sospensiva hanno a mio parere dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che questo provvedimento apporta delle lesioni irrimediabili al codice di procedura penale e all'articolo 111 della Costituzione, che vigila sulla ragionevole durata del processo

farlo in questo brusìo. Per cortesia. PARDI *(IdV)*. Il provvedimento è giunto in quest'Aula irrimediabilmente stravolto rispetto alla sua premessa costitutiva tramite emendamenti inammissibili secondo l'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato. Questo provvedimento si chiamava per il nome della prima firmataria Lussana. Se la collega Lussana della Camera avesse la fermezza d'animo del collega Cirielli rispetto ad avventure precedenti, forse chiederebbe che questo provvedimento d'ora in poi si chiami *ex* Lussana, perché così come esce non ha più nulla a che vedere con il testo originario. Di fatto, il testo di questo provvedimento tradisce in modo ipocrita, ma definitivo il suo stesso titolo. Il tema fondamentale della legge è accantonato e se ne introduce uno che ha un obiettivo molto chiaro e inequivocabile. La modifica degli articoli 190, 238-*bis*, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale determina degli effetti di questa natura. Si stabilisce che possono essere ammesse delle prove superflue, e questo costituisce una lesione all'autonomia della magistratura; si stabilisce che si può operare una dilatazione virtualmente infinita delle liste testimoniali, e questo incide ancora una volta sull'autonomia delle decisioni del giudice, che non può intervenire sulla limitazione dell'allargamento delle liste testimoniali. In questa maniera, l'insieme dell'istituto probatorio passa dalla condizione di elemento funzionale per il fine primario, della ricerca della verità, alla condizione di elemento che ha una funzione esclusivamente dilatoria, confliggendo apertamente con l'articolo 111 della Costituzione. L'ampiezza temporale non è determinata e non è determinabile. Si preparano processi in cui si sa quando si comincia e non si sa quando si finirà, perché è imprevedibile l'ammissione di prove superflue e la dilatazione delle liste testimoniali. Ci sono ancora degli elementi peggiorativi: la compromissione dell'articolo 238-*bis* stabilisce di fatto l'impossibilità di riferirsi a sentenze passate in giudicato; si stabilisce la possibilità di esaminare di nuovo tutte le persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza. E poi c'è una firma che stabilisce con chiarezza qual è l'obiettivo finale di questa legge, quando si dice che tutto ciò che è stato detto si applica solo ai processi in cui non sia stata dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado. Con questo provvedimento andiamo incontro ad una combinazione schiacciante tra il processo lunghissimo, da una parte, e la prescrizione brevissima dall'altra. L'illustrazione sapiente che i colleghi hanno dedicato alle loro questioni pregiudiziali dimostra che dal punto di vista dei criteri generali questa legge è del tutto insensata. Non c'è motivazione al mondo per sostenere che in Italia ci sia bisogno di deturpare e distorcere all'origine, in modo costitutivo, il processo penale in questa maniera. C'è un solo motivo che regge questo bisogno: è la necessità di salvare dai processi il Presidente del Consiglio. con la sua azienda pochi giorni fa ha dovuto pagare 560 milioni di euro perché l'insieme dei dibattimenti che si sono svolti in merito hanno stabilito che l'azienda editoriale Mondadori era stata sottratta,

pagato da un dipendente del Presidente del Consiglio, nella persona dell'onorevole Previti, che è stato condannato per questo: condanna per corruzione in atti giudiziari, condanna per risarcimento danni. Viviamo in una situazione avvilente in cui il Presidente del Consiglio è l'utilizzatore finale di un'operazione di corruzione giudiziaria

perché mai, in qualsiasi altra democrazia occidentale, un individuo simile avrebbe potuto accedere alle Aule rappresentative e mai avrebbe potuto...

Se poi la maggioranza gode di questa sorta di pantano faccia pure. Purtroppo, il Parlamento italiano, le Assemblee rappresentative elette dal popolo sono le testimoni impotente di una condizione che in qualsiasi altro Paese democratico sarebbe stata impossibile. di quest'Aula, dopo aver fatto elogi sperticati e retorici all'atmosfera di collaborazione

cari colleghi della maggioranza, che in questo momento vi rifiutate di considerare la validità sostanziale del risultato che ha dimostrato che il popolo italiano non sopporta e non sopporterà le leggi *ad personam*, vi assumete una responsabilità pazzesca. Fatti vostri! Noi ve lo diciamo chiaramente. Voi siete di fronte alla possibile bocciatura, da parte della Corte costituzionale, di una legge che ha sei o sette profili di incostituzionalità e siete esposti di fronte alla possibilità di una nuova iniziativa referendaria che ricaccerà nel novero delle cose che non esistono non esistono questo provvedimento insensato. Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'articolo 97 del Regolamento del Senato recita al suo primo comma: "sono improponibili... emendamenti... che siano estranei all'oggetto della discussione." La discussione di questo disegno di legge verte sulla inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Mi chiedo cosa c'entri con questo oggetto la non ammissibilità dei testimoni in ogni procedimento. Credo che qualsiasi persona di buon senso, che conosca anche la lingua italiana e che pure non abbia una particolare competenza in materie giuridiche, si renda conto che vi è totale estraneità di materia. vi è una netta contraddizione con l'articolo 97, comma 1, del nostro Regolamento; mi domando dunque per quale motivo sia stato consentito un emendamento di questo tipo. Poi c'è un altro profilo credo molto importante. Abbiamo sempre detto - lo ha detto questo Governo e questa maggioranza

delle norme e delle riforme. Ora, non c'è alcuna ragione di introdurre una norma di questo tipo, che, abbiamo sottolineato, fra l'altro si inserisce in un contesto del tutto ultroneo.

a individuare i colpevoli di determinati procedimenti era uno dei *must*, uno degli obiettivi... Chiedo, in particolare agli amici della ex Alleanza Nazionale,

Signora Presidente, è vero: le opposizioni hanno presentato undici questioni pregiudiziali e una questione sospensiva; il Gruppo del Partito Democratico ha presentato nove questioni pregiudiziali e una questione sospensiva. Poco fa, il presidente Schifani ha affermato, fra l'altro, che il numero delle questioni pregiudiziali offerte all'attenzione dell'Aula del Senato costituisce un fatto eccezionale rispetto alla prassi di quest'Aula. È vero, signora Presidente: abbiamo presentato il giusto numero di questioni all'altezza di questa seduta, una seduta tutta all'insegna dell'orgoglio - il vostro irriducibile pregiudiziali - le nostre - avverso l'impianto di un provvedimento, anch'esso sì, eccezionale; forse troppo eccezionale. Per obbligare il Senato a discutere di un testo tanto irriducibile quanto assurdo avete violato le norme che regolano l'esercizio del più alto dei poteri che si esercitano in democrazia: il potere legislativo esercitato dal Parlamento.

della maggioranza).* Mi piacerebbe che qualcuno di voi, soprattutto quelli non presenti nella scorsa legislatura, si andasse a leggere qualche passaggio di atti parlamentari, quando presentavate alcune questioni pregiudiziali che non avevano né capo né coda, prima di fare commenti nell'ambito di quest'Aula.

l'approvazione di un provvedimento che non è funzionale e che nulla apporterà di positivo al sistema del processo penale. non c'è bisogno che le opposizioni si adoperino per impedire l'approvazione di questo inguardabile disegno di legge, perché sono mesi ormai

il 2.0.200 -, dopo aver armonizzato i tempi della discussione, signora Presidente. Insomma, prima avete provato a tapparci la bocca contingentando i tempi e poi fate le proposte di merito. Diteci voi se questo è esercizio della democrazia. grazie a questa legittima protesta che il Presidente del Senato, poco fa, ha revocato questa armonizzazione,

Forse, signora Presidente, le truppe sono stanche e hanno bisogno, dopo tutte queste battaglie, di riprendere un po' di fiato. Il provvedimento che oggi è qui in Aula è qui in Aula è totalmente diverso da quello licenziato dalla Camera, e voi lo sapete, perché la Camera l'ha licenziato il 17 febbraio 2011, e noi siamo qui a parlare di un testo completamente diverso. L'emendamento del collega Mugnai, che sta molto attento ad ascoltare e - lo so - é molto bravo, ha introdotto un tema estraneo - ecco perché è bravo - e lo ha introdotto bene, ma non c'entra niente con il provvedimento licenziato dalla Camera il 17 febbraio.

La profonda modifica del contenuto normativo di questo disegno di legge all'attenzione dell'Aula è cosa completamente diversa da come veniva rubricato una volta licenziato dalla Camera dei deputati. Lei, omette - ecco il piccolo limite, che ovviamente è scientifico e fatto *cum grano salis* da parte sua - il fatto che nel disegno di legge non si parla né di rito abbreviato né di ergastolo. Il titolo di questo disegno di legge non esiste nel contenuto del disegno di legge stesso. Ora, noi possiamo far finta di non vedere, ma è difficile che gli italiani continuino a fare lo stesso. Queste modifiche escludono principalmente, signora Presidente, il vaglio del giudice in ordine all'eventuale carattere manifestamente superfluo e rilevante della prova. Mi verrebbe da dire, in modo poco elegante, collega Mugnai, e lo dico a lei per colleganza professionale: quanti studi legali saltano di gioia il giorno dopo che questo disegno di legge diventa legge di questo Paese e parte dell'ordinamento giudiziario? Soprattutto, quanti studi penalistici studi penalistici sono contenti del risultato che deriverebbe da questo provvedimento? Non lo devo certo spiegare, perché c'è qualcuno che in modo più appropriato di me lo ha fatto. Presidente, questi effetti dilatori appaiono ancora più gravi ove si consideri che, in base al comma 5 dell'articolo 1, la disciplina si applica anche ai processi in corso, e perché togliersi questa soddisfazione di non modificare le regole del gioco mentre il gioco è in corso, collega Mugnai? Come si fa, per per una volta, a far finta che i processi terminino con le regole con cui sono iniziati e i nuovi inizino con quelle che il legislatore poi approva? È troppo difficile usare questa tecnica, che è normale, e quindi, evidentemente, evidentemente, se non si accoglie l'idea di far decorrere la nuova normativa con i nuovi processi, c'è qualche piccolo processo in corso sul quale volete intervenire. Ovviamente a pensare male si fa sempre bene, come diceva qualcuno più autorevole di me, però potremmo anche sbagliarci. Appare evidente

forse si applicano al Presidente del Consiglio dei ministri. Non lo so. Lo verificheremo in corso d'opera quando, una volta che questo disegno di legge sarà diventato legge dello Stato,

Presidente, sarebbe molto interessante se lo stesso collega Mugnai, per conto della maggioranza, provvedesse ad un testo corretto dell'emendamento presentato in Commissione dove, ad esempio, risolvesse i problemi per i processi in corso (già sarebbe interessante), oppure parlasse dell'irrilevanza delle prove sottoposte al vaglio del giudice o della strumentalità di un'azione difensiva che serve ad altro e non certo a dichiarare il giusto processo. Riteniamo che ci siano fondate ragioni - molto fondate - per pensare che l'ipotesi normativa che introduce

di quelle che subiscono, delle parti lese, delle parti civili, delle persone offese dal reato, che saranno totalmente prive di qualsiasi forma di difesa grazie a questo vostro provvedimento. *(Applausi

alcuni componenti del Consiglio superiore della magistratura, di fatto intervenendo e interferendo sul processo di approvazione che questo ramo del Parlamento sta conducendo in ordine al provvedimento esame, si sono espressi, manifestando stupore e scandalo, affermando che viene introdotta la inedita facoltà per l'imputato di interrogare personalmente i soggetti che lo accusano, e non già solo attraverso il proprio difensore.

nell'alveo di ciò di cui realmente dovremmo parlare, al di là di strumentalizzazioni e di chiavi di lettura assolutamente improprie. È sufficiente una lettura del testo dell'articolo 111 della Costituzione, per come lo stesso attualmente recita, per rendersi conto che la persona imputata

Ho voluto dire questo perché credo che nell'esame delle questioni pregiudiziali e sospensive non si possa prescindere da una serie di considerazioni di carattere preliminare, per poi arrivare a quelli che sono sostanzialmente i due motivi fondanti sulle quali sono state incernierate. Intanto, consentitemi di dire che questo non è il testo di chi vi parla, ma è quello licenziato dalla 2a Commissione permanente del Senato, sia pur a maggioranza, quindi evidentemente già attraverso una prima delibazione. Il testo, per come oggi si presenta all'esame del Senato, nella parte modificativa dell'originale impianto in tema di rito abbreviato, licenziato dalla Camera dei deputati, è tale avendo il relatore recepito espressamente ciò che in sede di audizioni la stessa Associazione nazionale magistrati aveva prospettato, ovverosia il fatto l'eventuale meccanismo che si voleva introdurre non poteva che collocarsi a valle del procedimento, e non a monte, e quindi con riferimento alla sanzione erogata in concreto e non alla facoltà che chiunque ha di poter adire il giudizio abbreviato.

Il titolo I del libro terzo del codice di procedura penale, quello in cui è inserito in modo sistematico l'articolo 190, recita: «Disposizioni generali», e si riferisce agli istituti nella loro ontologica, individuale accezione; tant'è che a partire dal successivo titolo II si disciplinano i vari mezzi di prova: la testimonianza, l'ispezione, la ricognizione e quant'altro.

tant'è che arriviamo a dire che, laddove in concreto si vuole irrogare la sanzione dell'ergastolo non si potranno più utilizzare le diminuenti del rito; *ergo*, con riferimento all'abbreviato condizionato, va da sé che necessariamente si imponeva un attento esame ed una eventuale revisione del meccanismo attraverso il quale si forma la prova in contraddittorio tra le parti, come previsto all'articolo 111, salvo altrimenti non andare ad introdurre una precisa violazione del diritto di difesa.

quello del 1989 a firma Pisapia ed altri. Sappiamo perfettamente infatti che la parte civile nell'attuale processo penale ha un ruolo diverso. E' bene ricordare che la parte civile, nell'attuale codice di rito, non può impugnare la sentenza se non per i soli effetti civili. Svolge attività diverse sino al momento in cui è solo persona offesa, ma quest'altro aspetto, proprio riferendosi alla parte civile, parla di fatti che ineriscono anche quelli che sono i profili poi legati al risarcimento del danno. Inerente e pertinente sono assolutamente sinonimi. il problema fondamentale. Qui si sta semplicemente cambiando il criterio di valutazione, passando da un mero giudizio, che può essere anche apodittico in termini di rilevanza, ad un giudizio di carattere pertinente, cioè attinente al fatto, in ossequio al disposto dell'articolo 111 della Costituzione. Ma questo è stato già detto. E così, parlando di pertinenza si potrà quindi indicare sterminate liste testimoniali, si potranno portare come testi tutti coloro che hanno visto la partita di calcio, e quant'altro. Onorevoli colleghi, chi lo dice non ha letto le norme del codice di rito. L'articolo 468 del codice di procedura penale, quello che dà il potere di ridurre le liste manifestamente sovrabbondanti, non è toccato! Cambia semplicemente il criterio attraverso il quale quelle liste saranno formate, ricordando sempre che la prova, intesa come mezzo di prova, è un *unicum*. E ugualmente rimane l'altro filtro, l'articolo 495, cioè quello che nel dibattimento riconosce al giudice il potere di revocare i mezzi di prova manifestamente superflui.

che il mezzo di prova deve essere pertinente e, quindi, non potrà mai essere né manifestamente superfluo né irrilevante, senatore Carofiglio, che con grande suggestione ha evocato questo! Perché ciò che è pertinente fatalmente non è né superfluo né irrilevante!

Senatore Mugnai, come ad altri colleghi ho concesso anche a lei del tempo ulteriore.

che questo provvedimento è arrivato al Senato con un titolo e un contenuto totalmente diverso da quello oggi al nostro esame.

e con il titolo del provvedimento stesso. Delle due l'una, signor Presidente: o gli effetti delle norme che si vogliono qui introdurre modificando il codice di procedura penale sono quelli che tutte le opposizioni denunciano, denunciano, cioè quelli di attribuire alle difese degli imputati sostanzialmente la possibilità di non fare processi, perché si potranno richiedere le liste testimoniali smisurate,

direttamente, oppure il provvedimento ha il contenuto di cui parlava il senatore Mugnai, oppure ci sarà un'altra interpretazione. Ora, poiché, signor Presidente - caso unico

di essere presente in Aula, anche perché è senatore e quindi non gli dovrebbe essere difficile, per partecipare alla discussione di questo provvedimento e, almeno domani in sede di replica, di farci conoscere l'opinione del Governo, e la sua, su un provvedimento come questo, che potrebbe definitivamente disastrare la giustizia penale italiana.

di consentire alla senatrice Della Monica di svolgere il suo intervento.

seduta. Comprendo che ogni volta che si parla di giustizia ordinaria, cercando di riportare il discorso sull'efficienza della giustizia, non interessa a nessuno. E questo è un concetto che mi è chiarissimo.

*(PD)*. Ricomincio da capo. Il disegno di legge che oggi è all'esame dell'Aula del Senato, e che vedeva come prima firmataria l'onorevole Lussana, escludeva per i reati puniti con l'ergastolo l'applicazione dei benefici previsti per il rito abbreviato. Aveva quindi come unico obiettivo un maggior rigore punitivo nei processi per gravi reati. È intervenuta poi una riscrittura del regime processuale sulla prova, del tutta estranea all'originario intento, che ha la finalità di rallentare a dismisura la durata di tutti i processi penali attualmente in corso, con l'eccezione - guarda caso - per quelli per cui sia stato già chiuso il dibattimento di primo grado. Le disposizioni di maggiore interesse che ora esaminerò riguardano la modifica degli articoli 190, 495 e 238-*bis* del codice di procedura penale, che disciplinano l'esercizio del diritto alla prova e l'acquisizione probatoria. Ovviamente, per comprendere la portata di queste disposizioni, bisogna effettuare un confronto tra la normativa esistente e quella proposta, confronto che al momento vi risparmio, poiché è ben evidenziato per iscritto.

Capisco che debbano difendere una legge indifendibile, ma non si possono prendere in giro i cittadini italiani. La nuova formulazione dell'articolo 190 del codice di procedura penale presenta infatti degli effetti devastanti per l'economia processuale, e questo al di là del giudizio abbreviato, che finisce per vedere totalmente svilita la propria natura di giudizio allo stato degli atti che collega la diminuzione di pena a ragioni di economia processuale che presiedono il rito. ragioni per cui questa nuova formulazione ha effetti devastanti sono le seguenti. Innanzitutto viene introdotta come principio generale una sanzione di nullità prima inesistente, addirittura relativa alla fase di ammissione delle prove, il che finisce per innescare un pericoloso cancro nella tenuta dei processi. É appena il caso di ricordare che il sistema processuale è fondato sul principio della tassatività delle nullità proprio per evitare problemi simili che porterebbero ad una infinita serie di annullamenti delle sentenze. Il secondo punto è che il sistema raggiunge il culmine della sua pericolosità allorquando il potere attuale del giudice di escludere le prove vietate dalla legge e quelle che sono manifestamente superflue e irrilevanti viene sostituito con l'obbligo di ammettere le prove, ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. del problema sta proprio in questo, ossia nel passaggio dalle prove superflue o irrilevanti a quelle manifestamente non pertinenti. L'attuale disposizione, infatti, è finalizzata ad un principio di economia processuale potendo essere superfluo e irrilevante qualcosa che serve a dimostrare ciò ciò che è stato già sufficientemente provato, mentre il concetto di non pertinenza è qualcosa di ben diverso, perché riguarda più in generale il legame tra il fatto il senatore Mugnai provi un senso di fastidio quando io parlo dell'accoltellamento allo stadio per cui, invece di sentire tre testimoni che sono in grado di riferire il fatto oppure di guardare il filmato che è stato fatto dalle forze di polizia, dobbiamo magari sentire 80.0000 testimoni. Ma l'effetto devastante è è questo. Non ci prendiamo in giro. In detta situazione si cerca quindi di introdurre nel nostro ordinamento una specie di diritto potestativo insindacabile alla prova, escludendo che il giudice possa valutare la natura manifestamente superflua o irrilevante delle prove richieste, e quindi gestire l'andamento del processo in funzione di un accertamento processuale che si svolga secondo i canoni costituzionali della ragionevole durata, ma anzi imponendo di fatto una ammissione di qualsiasi prova che non risulti manifestamente non pertinente, e dunque non estranea al *thema* *decidendum*. La norma ha lo scopo di consentire ai difensori di dilungare *ad libitum* la durata dei processi peraltro ben conosciuta in alcuni "noti" processi - e se il tutto fosse coordinato con la prescrizione breve, per parafrasare il titolo di un film, si sarebbe creata la tempesta perfetta. Il Consiglio superiore della magistratura ha già dato un parere, poiché queste norme erano inserite nel disegno di legge governativo n. il parere del 23 luglio 2009 - tanto vituperato, di organo che è chiamato ad occuparsi della ricaduta in ambito giudiziario delle leggi che il Parlamento approva - era che che «La soluzione normativa indicata determina una irragionevole delimitazione della discrezionalità connessa all'esercizio della funzione giudicante e un pesante limite al celere svolgimento del giudizio (...)». Guarda Guarda caso, questa valutazione coincideva con quella degli avvocati dell'Unione camere penali, che aveva espresso sul punto notevoli perplessità. E questo è più che comprensibile, perché sostanzialmente si consacra un diritto all'abuso processuale, legittimando tutte le tattiche processuali dilatorie, comprese le impugnazioni pretestuose allo scopo di ottenere l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Colleghi della Lega, la sicurezza di questo Paese va a

È vero che tale disposizione ricopia il testo del comma 3 dell'articolo 111 della Costituzione, ma la facoltà per l'imputato di interrogare personalmente i soggetti che lo accusano, non più solo attraverso il proprio difensore, ha una potenzialità intimidatoria sul teste o sul collaboratore di giustizia inopportuna, inaccettabile, irragionevole, al di là di una regolamentazione di una facoltà, che può risolversi, in assenza di una regolamentazione, in un abuso. Voi immaginate Totò Riina che interroga i collaboratori di giustizia o i testimoni o qualcuno in Aula? Ve lo immaginate? È questo che si vuole?

ancora più rigorosi i limiti imposti al giudice dibattimentale il quale - a causa dell'"e" da leggersi come "*and*" e non certo come alternativa e del successivo "salvo che" potrà revocare l'ammissione solo delle prove di prove che presentino congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche: a) siano superflue; b) siano manifestamente non pertinenti (oltretutto ciò che è manifestamente non pertinente già da sé e anche superfluo, ma la lingua c) non siano state richieste a prova contraria di prove già assunte. **In conclusione**: siamo ai limiti della follia giuridica (forse solo sul set della trasmissione "Scherzi a parte"), in quanto sfido chiunque a trovare casi in cui si verificano contestualmente le tre indicate indicate condizioni, con la conseguenza che il giudice di fatto sarà in ostaggio delle prove richieste dalle parti che determineranno in tal modo (sempre con la spada di Damocle della nullità in caso di rigetto) i tempi del processo quantomeno fino alla sua prescrizione. È questo che si vuole: distruggere la giustizia penale, in danno dei cittadini. Ciò a tacere che, in conseguenza della modifica proposta sul terzo comma dell'articolo 190, non sarebbe neppure possibile per il giudice intervenire in un secondo momento, con la revoca delle prove ammesse, malgrado sia divenuta evidente la sopravvenuta superfluità di ulteriori assunzioni di testi o collaboratori, in seguito all'istruttoria dibattimentale svolta. del codice di procedura penale. La modifica proposta fa cadere l'ultimo baluardo di possibile resistenza alla durata dei processi. La norma significa che «anche se la sentenza è irrevocabile il processo è sostanzialmente da rifare». È questo che volete? Facciamo un esempio a caso: cosa accade per il processo Mills? La risposta è, ovviamente: lo rifacciamo tutto. Si guardi bene, la norma è infida, perché imponendo sostanzialmente il rifacimento del processo, consente di attaccare «il fatto accertato» (comma 1) nella sentenza irrevocabile, con la conseguenza che qui non si parla di prova di responsabilità del soggetto, ma addirittura di rifare la prova (orale) circa l'esistenza del fatto. Per essere chiari, le sentenze irrevocabili si potrebbero continuare ad acquisire, ma tutta l'istruttoria dibattimentale già svolta nei relativi processi, sulla base della semplice richiesta dell'imputato dovrebbe essere necessariamente interamente ripetuta. Si tratta di una previsione contraddittoria ed irragionevole, poiché se si consente l'acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova dei fatti accertati e questo accertamento rimane definitivo in mancanza di una richiesta dell'imputato, non si comprende perché sia imposto di svolgere nuovamente un'istruttoria sugli stessi fatti, solo che l'imputato lo richieda. O c'è un giudicato o non c'è. Ed è evidente che l'esclusione, in questo caso, di un adeguato filtro selettivo sull'acquisizione probatoria da parte del giudice altro non farebbe che determinare un ulteriore abnorme prolungamento dei tempi del dibattimento penale. conclusione: tornando all'esempio a caso fatto prima in un processo come quello Mills, bisognerebbe (quantomeno fino alla maturazione della prescrizione breve) provare non solo la responsabilità dell'attuale imputato, (cosa assolutamente rispondente a diritto) ma anche ritornare a provare l'esistenza del fatto posto alla base di tale responsabilità. La domanda sarebbe: vi fu una falsa testimonianza, accertata con sentenza passata in giudicato a carico di Mills?

per inserire un testo sbilenco, di difficile lettura ed interpretazione. Infatti, se da un lato si introduce il riferimento all'articolo 190 del codice di procedura penale, ovviamente nel testo modificato nel suo complesso, e conseguentemente il riferimento sia alla possibilità di esercitare la «facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore», sia alla sanzione di nullità in caso di mancata ammissione di prove pertinenti, dall'altro si aggiunge il sibillino inciso «in quanto applicabile». Dunque, si applica o non si applica il processo abbreviato? Il tutto diventa ancora più complicato dato che si lascia vivere l'inciso "se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili". Al riguardo il giudice sembra chiuso in una forbice tra il rispetto della natura del giudizio ("abbreviato", per l'appunto) e la sanzione di nullità, e ciò finisce per vanificare la strada che la Corte di cassazione aveva sapientemente tracciato allorquando aveva affermato che il legislatore, attraverso l'utilizzazione dell'espressione "integrazione" probatoria, ha evidentemente voluto escludere la possibilità che la richiesta di essere giudicati con le forme del rito abbreviato possa essere subordinata alla mera riproposizione con le forme del contraddittorio (ancorché in un'ottica di possibili precisazioni) di elementi probatori già raccolti nella fase delle indagini preliminari.

ponendosi, siccome circoscritte e strumentali, ai fini della decisione di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa e dall'altro che, per l'identificazione del carattere di necessità dell'integrazione probatoria richiesta, deve farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'articolo 190, comma 1, del codice di rito. La proposta di legge che giunge oggi in aula, stravolgendo il testo originario del disegno di legge proposto dalla Lega e approvato alla Camera dei deputati è per la giustizia la minaccia di una tragedia ancora maggiore, se possibile, della prescrizione breve, che inciderebbe "solo" , si fa per dire, sui processi agli incensurati, già favoriti dalla sciagurata legge ex-Cirielli del 2005. Il cosiddetto processo lungo, processo lungo, se approvato, sarebbe un incentivo a giovarsi della prescrizione e per questo a moltiplicare tecniche dilatorie e impugnazioni infondate; tutti imputati recidivi o incensurati avrebbero interesse a rallentare ovvero a paralizzare la giustizia penale, per la cui efficienza e celerità questo Governo nulla ha fatto e nulla vuol fare: si ridimensionerebbe perfino l'interesse a definire il processo, patteggiando la pena. E il rito abbreviato, prolungabile anch'esso con tecniche dilatorie, consentirebbe solo un ingiustificata riduzione di un terzo della pena,

questo non può certo avvenire favorendone l'estinzione, con diniego di giustizia per le parti offese e clamorosa rinunzia alla tutela della sicurezza dei cittadini. La finalità della normativa è semplicemente quella di favorire una persona, il Presidente del Consiglio, per salvaguardarlo dai processi

alcune delle disposizioni più significative, integrando l'elenco che ho proposto questa mattina illustrando la questione pregiudiziale: • Legge sulle rogatorie internazionali (legge n. 367 del 2001): limitazione dell'utilizzabilità delle prove acquisite attraverso una rogatoria (trova applicazione anche al processo "Sme-Ariosto 1" per corruzione in atti giudiziari). • Depenalizzazione del falso in bilancio (legge n. 61 del 2002): modifica della disciplina del falso in bilancio (nei processi "All Iberian 2" e "Sme-Ariosto2" Berlusconi viene assolto perché "il fatto non è più previsto dalla legge come reato"). • "Legge Cirami" (legge n. 248 del 2002): introduzione fra le cause di ricusazione e trasferimento del processo del "legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice" (la norma utilizzata per spostare il processo da Milano a Brescia non ottenne, però, i risultati sperati). non ottenne, però, i risultati sperati). • "Lodo Schifani" (legge n. 140 del 2003): introduzione del divieto di sottoposizione a processo delle cinque più alte cariche dello Stato tra le quali il Presidente del Consiglio in carica, dichiarata incostituzionale dopo pochi mesi, con sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004. Condono edilizio nelle aree protette (legge n. 308 del 2004): estensione del condono edilizio alle zone protette (comprensiva la villa "La Certosa" di proprietà di Berlusconi). "Legge ex Cirielli" (legge n. 251 del 2005): riduzione dei termini della prescrizione (denominata anche legge salva-Previti, ha introdotto una riduzione dei termini di prescrizione per gli incensurati e trasformato in arresti domiciliari la detenzione per gli ultrasettantenni, con ripercussioni rispetto ai processi "Diritti e"MiIls" a carico di Berlusconi). • "Legge Pecorella" (legge n. 46 del 2006): introduzione dell'inappellabilità da parte del PM delle sentenze di proscioglimento, dichiarata incostituzionale dopo pochi mesi, con sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007. "Lodo Alfano" (legge n. 124 del 2008): introduzione di un nuovo divieto di sottoposizione a processo delle quattro più alte cariche dello Stato tra le quali il Presidente del Consiglio in carica, dichiarata incostituzionale dopo un anno, con sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009, per violazione degli

del giugno 2011. Di fronte a obbrobri giuridici come quelli sopra elencati, di fronte a norme che violano ed eludono i principi costituzionali di eguaglianza, di ragionevolezza, di ragionevole durata del processo, quali quelle inserite a sorpresa nell'Atto Senato n. 2567, non si può che rimanere sbigottiti. Colleghi della Lega e del Popolo della Libertà, ma quale democrazia volete per questo Paese, quale giustizia, quale sicurezza?!

il tempo d'intervento dei singoli colleghi è solo segnalato alla Presidenza, non è tassativo, evidentemente. Tuttavia, per consentire una migliore organizzazione dei lavori posso immaginare che

In particolare, me lo consentiranno i colleghi dell'opposizione, a quei pochi colleghi della maggioranza che sono in Aula: vuol dire che ha qualcuno interessa ancora il tema della giustizia e anche sentire qualche considerazione critica da parte dell'opposizione. In questi ultimi tempi mi sono interrogato a più riprese sul perché di questa incessante ondata di impopolarità della politica, questo distacco della gente, dei cittadini da tutti noi; sul perché si è alzato un muro tra la realtà di tutti i giorni e il nostro mondo.

lontani dai bisogni della gente, lontani dal 30 per cento di giovani che non hanno e non avranno lavoro, lontani dal mondo del precariato, lontani quindi da tutti questi problemi che dovrebbero essere affrontati con ben altra grinta e velocità in queste Aule, lontani da tutti,

Ed è triste che questa ondata di impopolarità, che viene quasi esclusivamente dalle vostre responsabilità, finisca poi per travolgere tutti noi, schiacciati da una logica di Parlamento che fa tremare i polsi:

-ignorano totalmente l'espressione popolare e i recentissimi risultati referendari, che pur hanno ricordato al Governo, al*Premier* in particolare, e alla maggioranza come i cittadini siano stufi di assistere ai continui tentativi di introdurre leggi *ad personam*. Ebbene, il provvedimento che oggi questa Aula è chiamata in tutta fretta - chissà perché poi questa fretta - ad affrontare e rispetto al quale ci dichiariamo fortemente contrari si colloca proprio in quest'ottica. Dicevo in tutta fretta, nonostante la richiesta delle opposizioni, compatte su pregiudiziali e sospensive e su inversioni dell'ordine del giorno. In tutta fretta perché? perché? Abbiamo chiesto di trattare innanzi tutto un decreto che prevede 18 mesi di carcerazione - come la vogliamo chiamare? - per chi non per chi non ha commesso alcun reato. Discutiamo di questo, della libertà della gente. Ma come si giustifica questa fretta se non con una prova muscolare? E si giustifica? Esiste il voto di scambio, ma qui in Parlamento si è inventato un istituto nuovo che si chiama provvedimento di scambio. Il provvedimento di scambio all'interno della maggioranza: io ti do questo e tu mi dai questo. Parlavo di *escamotage*, di stratagemmi. Sappiamo che il testo in esame nasce in origine per modificare le previsioni che regolano il cosiddetto giudizio abbreviato, allo scopo di evitare l'applicabilità del rito speciale e dei relativi benefici ai delitti più gravi puniti con l'ergastolo: un testo del tutto rispettabile. Ma quello che abbiamo di fronte è tutt'altra cosa, un provvedimento molto lontano dall'intento originario. Il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato, di cui faccio parte, ha stravolto quasi completamente l'impianto normativo iniziale, intervenendo fortemente sul regime di acquisizione delle prove. Dio non voglia che io sia mai imputato, ma se dovessi esserlo un giorno, cercherei in tutti i modi di farmi

In buona sostanza, si è apportata una modifica che interviene in materia di riforma del codice di procedura penale, in particolare rispetto al regime delle prove, all'interno di un testo che aveva come oggetto l'inapplicabilità del rito speciale ai delitti puniti con l'ergastolo. Approfondendo il testo, che è già stato approfondito in maniera straordinaria da chi mi ha preceduto, in particolare da Silvia Della Monica, ci si ci si accorge poi di quanto questo presenti tratti di evidente incostituzionalità. La versione licenziata dalla Commissione giustizia modifica in maniera grossolana alcune norme del codice di procedura penale relative non solo ai presupposti stessi del giudizio abbreviato, ma anche al diritto di prova, ai provvedimenti del giudice in ordine alle prove, alle sentenze irrevocabili e, infine, alle decisioni del giudice sul giudizio abbreviato. L'obiettivo ultimo di tale progetto e di tutte queste modifiche non sfugge a nessuno: si tenta con esso di bloccare la giustizia penale anziché alleggerirla, come più volte proclamato da questa maggioranza, provando Siamo di fronte a una forma di schizofrenia, perché dapprima il Governo propone il cosiddetto processo breve, propagandando la necessità di sollevare quel macigno rappresentato dalla lunghezza dei tempi della giustizia e presentando tale lentezza come un ulteriore freno all'economia del nostro Paese e poi, per contro, presenta a questa Aula e al Paese un provvedimento che dilata in modo indiscriminato ogni processo. Si tratta di un disegno di legge che presenta un'ulteriore anomalia: aumentando le potestà dell'imputato finisce per svilire il ruolo del giudice quale *dominus* del processo, in assoluto dispregio anche di altre figure determinanti quali il pubblico ministero o la persona offesa. Il presidente Schifani proprio oggi ha parlato della magistratura come un baluardo della legalità; ma non ci prendete in giro: voi disprezzate la magistratura, la temete e la delegittimate. Il provvedimento in discussione si pone in aperto contrasto soprattutto con la nostra Costituzione che, all'articolo 111, quello che ha ricordato il collega Mugnai, recita «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato della legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità... La legge ne assicura la ragionevole durata». Parliamo, dunque, di giusto processo, ragionevole durata e contraddittorio tra le parti in condizioni di parità. Basta esaminare il testo per accorgersi di come questo disattenda ognuno di questi elementi. È indubbia prima di tutto la totale mancanza di parità tra le parti, dal momento che le novelle che si intendono introdurre dimostrano di considerare l'imputato come il nuovo vero *dominus* del processo e tutti gli altri soggetti come elementi accessori. Si intende così sancire un vero e proprio processo dell'imputato, trasformando la fase dell'istruzione dibattimentale da strumento utile alla ricerca delle verità in nuovo sotterfugio per estendere i tempi processuali in vista di un'auspicata prescrizione. Tale intento è ancora più chiaro se si analizza la modifica degli articoli 190 e 495. Il primo è relativo al diritto di prova, stravolto dal presente disegno di legge. PRESIDENTE.

*(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Si inserisce il diritto potestativo per l'imputato di interrogare o far interrogare chiunque renda dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione nonché l'interrogatorio di persone a sua difesa alle condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Ad ogni imputato basterà indicare nella propria lista testimoniale centinaia di testimoni, anche solo lontanamente attinente ai fatti. La collega Della Monica ha fatto l'esempio dello stadio. ho uno più significativo e più bello, a mio avviso. Prendiamo un imputato di sfruttamento della prostituzione minorile: quante prostitute potranno essere chiamate all'interno di un processo? Tutte. Se fossi l'avvocato le chiamerei tutte, perché tutte possono dirci qualcosa, guai a dire che sono poco attinenti al processo! Tutto questo - è chiaro - condurrà a due risultati: prolungare a dismisura ogni processo e provocare un indiscriminato aumento delle dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione. L'altra prevista modifica relativa all'articolo 495 riguarda i provvedimenti del giudice in merito alla prova del dibattimento. Con il nuovo testo si arriva perfino a escludere la revocabilità delle un'ulteriore prova di come si legittimi e autorizzi una serie di inutili attività purché volute dall'imputato. Ancora una volta, si preferisce la dilazione dei tempi processuali all'efficienza della giustizia, contravvenendo a quanto prescrittoci reiteratamente dagli organi giurisdizionali europei, che continuano a condannarci per l'eccessiva lunghezza dei tempi delle procedure giudiziarie e penali. Un intento perseguito anche mediante un ulteriore tassello, forse il più bello di tutti, che modifica persino la cosiddetta *res iudicata*. Se oggi, infatti, si permette l'acquisizione al processo di sentenze irrevocabili passate in giudicato, secondo il nuovo testo le parti potranno ottenere l'esame anche delle persone le cui dichiarazioni sono state già utilizzate per le motivazioni della sentenza. individuare un esempio calzante. Prendiamo, a caso, il processo Mills: quante persone già interrogate in quella sentenza passata in giudicato potranno essere di nuovo chiamate fino ad arrivare alla prescrizione? Ognuna di queste modifiche si applicherebbe ai processi in corso per i quali non sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado, con l'effetto di congestionare il processo con una serie di attività con una serie di attività istruttorie anche superflue, rimesse all'indiscriminata volontà dell'imputato, dilatando i tempi in violazione del principio della ragionevole durata del processo. Si tratterebbe di Si tratterebbe di un danneggiamento dell'intero sistema giudiziario in favore, ancora una volta, di interessi puramente personalistici, cui il mio Gruppo si oppone fortemente esprimendo, per ognuna delle ragioni suddette, totale contrarietà al provvedimento in esame.

il disegno di legge che oggi esaminiamo nell'Aula del Senato ha un titolo molto preciso: «Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo». Vorrei ricordare che questo disegno di legge, che arriva dalla Camera dei deputati, portava e porta tuttora la firma anche del Presidente del mio partito, l'onorevole Di Pietro,

L'articolato di questo disegno di legge, infatti, era assolutamente coerente con l'intitolazione che vi ho ricordato. I lavori della Commissione, però, come è già stato ricordato in più interventi, ci hanno consegnato un testo assolutamente, non solo stravolto, ma inaccettabile.

Questo comma, come l'Assemblea sa, è frutto dell'emendamento del senatore Mugnai. Questo emendamento - e quindi il comma che è stato introdotto nel testo del disegno di legge non ha niente a che vedere con l'impianto normativo che era uscito dalla Camera dei deputati e legittima il forte sospetto (poi vedremo perché)

infatti di introdurre una modifica all'articolo 238*-bis* del codice di procedura penale. Questa norma, nella sua attuale formulazione, consente l'acquisizione di una sentenza divenuta irrevocabile in un altro procedimento ai fini della prova del fatto in essa accertato. Ciò ovviamente non comporta assolutamente (questo è sempre stato molto chiaro) per il giudice alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti, né tanto meno dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione della sentenza che viene acquisita. Da sempre si è ritenuto (e da sempre così è stato) che il giudice, dovendo correttamente fare le sue valutazioni anche in riferimento ad altri elementi, conservi integra l'autonomia e la libertà di formulazione di giudizio. Quindi, questa norma, l'articolo 238-*bis* per come è oggi nel nostro codice di procedura penale, non inficia minimamente il principio del libero convincimento del giudice. Come si vorrebbe modificare questa norma secondo l'emendamento Mugnai? Mantenendo l'acquisizione della sentenza passata in giudicato, ma, nello stesso tempo, consentendo alle parti di riesaminare le persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza nell'altro procedimento. Quindi, l'emendamento Mugnai sostanzialmente vorrebbe consentire di rifare (anche integralmente, perché no?)

grado. Sostanzialmente questa norma si potrà applicare ai processi che, pure iniziati, non si siano ancora conclusi in primo grado. Ho rinvenuto, e non credo di sbagliare,

cui già si parlava dell'articolo 238-*bis* con l'intenzione di riformarlo, ma dell'applicabilità della norma modificata ai giudizi in corso non vi era traccia. Siamo nel 2008, ad inizio legislatura. Per carità, si può sempre ripensare alle proprie posizioni, ma voglio sottolineare questa particolarità. I sostenitori di questa riscrittura della norma dicono che il principio del contraddittorio nel momento formativo della prova deve essere esaltato, nel rispetto di quanto previsto dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 111. Effettivamente nel nostro ordinamento l'impianto accusatorio del codice, la centralità della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, l'esigenza di una valutazione genuina ed autonoma dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice sono sicuramente pilastri del nostro processo penale.

Ma così non è e cerchiamo di vedere velocemente perché. L'articolo 111 della Costituzione - che ho richiamato, come i fautori della

che, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, la prova debba formarsi nel contraddittorio delle parti e in ogni caso deve essere assicurata all'imputato la facoltà di fare interrogare i testimoni che lo accusano. L'articolo 238-*bis* - lo voglio ricordare all'Aula, al relatore Mugnai e alla maggioranza che, ahimè, sicuramente approverà questo scempio - è già stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, proprio in riferimento all'articolo 111 della Costituzione. La nostra Corte nel 2009 (quindi abbastanza recentemente) ha ricordato che questa disposizione, introdotta dopo le stragi verificatisi in Sicilia per contrastare più efficacemente la criminalità rganizzata, si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in un altro giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale utile alla decisione. Sempre la Corte ha avuto modo di dire che questo non intacca il basilare principio per cui ogni giudice è tenuto a formare il proprio convincimento in base alle prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante. Quindi, sostanzialmente, la Corte costituzionale in questa sentenza del 2009 ci ha detto che l'acquisizione del dato probatorio contenuto nella sentenza irrevocabile non è è momento autonomo rispetto all'utilizzazione che se ne farà poi nel processo ricevente. Quindi, momenti distinti, ma non autonomi. D'altra parte, vi sono altre numerose disposizioni nel nostro codice di rito che prevedono l'acquisizione di dati probatori esterni, ne indicano le condizioni, la finalità, e quindi in questa direzione si è mossa la Corte costituzionale.

ha, ovviamente, non nel momento dell'acquisizione ma in quello successivo della valutazione e utilizzazione. Quindi, una volta che la sentenza irrevocabile è acquisita al processo, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere in contraddittorio e, dunque, non vi è alcun tipo di violazione della prerogativa e dei nostri principi costituzionali. D'altra parte, l'articolo 238-*bis* non è l'unica norma che consente l'acquisizione di una sentenza irrevocabile in un altro procedimento; vi è, per esempio, anche l'articolo 236 del codice di procedura penale, che consente di acquisire sentenze divenute irrevocabili, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa o anche per valutare la credibilità di un testimone.

forse è perché l'interesse che si sta perseguendo con la modifica dell'articolo 238-*bis* non è quello nobile di fornire ai cittadini strumenti processuali rispettosi dell'articolo 111 della Costituzione, bensì quello di fornire ad un unico cittadino che ne ha interesse lo strumento processuale per affossare il suo processo e sferrare alla giustizia, che già soffre per i tempi lunghi, l'ennesimo colpo, forse questa volta mortale? Per caso il cittadino a cui volete offrire l'ennesimo salvacondotto dai processi si chiama Silvio Berlusconi? Per caso il cittadino Berlusconi sta affrontando un processo penale in cui è stata acquisita una sentenza irrevocabile? Per caso è il processo Mills? Forse il processo Mills è ancora aperto nella fase del dibattimento di primo grado e, quindi, gli si potrà applicare la modifica dell'articolo 238-*bis*? E allora, come si dice, tre indizi fanno una prova e possiamo quindi affermare con ragionevole certezza che sia provato che questa norma la volete per Silvio Berlusconi. senatore Mugnai - che non è in Aula, ma leggerà poi il mio intervento nel Resoconto - vorrei chiedere di avere l'onestà intellettuale di ammettere che l'esigenza di rendere applicabile la norma ai processi in corso è nata anche per anche per il processo Mills, per il quale nel 2008, quando lei ebbe a firmare il disegno di legge che ho ricordato e dove quella applicabilità non c'era, neanche c'era l'esigenza di far morire il processo. So che lei non può spiegarlo agli italiani, ma noi dell'opposizione, noi come Gruppo dell'Italia dei Valori, cercheremo di spiegarlo il più chiaro possibile, perché ancora una volta è chiaro che vi state prestando approvare una legge non che rende i cittadini uguali davanti alla legge, ma che rende un cittadino più uguale degli altri. E vi prego: smettetela di riempirvi la bocca con «il rispetto della Costituzione»: voi non sapete cos'è il rispetto della Costituzione, sapete solo obbedire

Signora Presidente, a onor del vero, non ho mai sentito un esponente della maggioranza riempirsi la bocca con il rispetto della Costituzione. Ora questo non vuol dire che necessariamente le vadano contro, ma neanche voglio fare l'avvocato difensore di chi non è in Aula in questo momento. La senatrice Della Monica ha concluso il suo intervento con un catalogo di leggi *ad personam,* formulando una domanda retorica, e cioè: quale tipo di democrazia ritiene la maggioranza di voler proporre al Paese? Ecco, purtroppo, non appartengo né alla scuola di pensiero per cui tre indizi fanno una prova, né tanto meno a quella che affronta le questioni con domande retoriche. Noi siamo di fronte ad un regime di antidemocrazia, un regime in cui le istituzioni quotidianamente violano la propria legalità e in particolare, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, non si tratta di violazioni che vengono denunciate da alcune parti dell'opposizione, bensì che vengono certificate un giorno sì e uno no della Corte europea dei diritti umani, relativamente

abbiamo un numero di prescrizioni che all'anno tocca le 120.000; abbiamo le carceri strapiene non soltanto di quasi 70.000 persone, a fronte di una capienza di 42.000, ma di persone che vanno dentro per reati bagattellari, quindi molto spesso ci è stato detto in una audizione nella Commissione straordinaria diritti umani che è difficile trovare all'interno delle carceri italiane chi ha commesso reati per il patrimonio superiori ai 500 euro. In questo contesto noi ci troviamo ad agire, e credo che questo contesto occorra ricordarlo,

non starò qui ad appesantire la discussione con gli stessi argomenti - che riguardano pochissimi individui di questa Repubblica: uno in modo particolare, cioè il Presidente del Consiglio. Pertanto, se il calendario va comunque rispettato, allo stesso tempo sappiamo che ci sono criteri di opportunità politica dell'introduzione di un provvedimento legislativo piuttosto che un altro. Tra l'altro questa discussione avviene alla vigilia di quello che probabilmente negli ultimi anni o decenni si caratterizzerà per essere il più grande appuntamento di riflessione e di proposta relativamente all'amministrazione della giustizia, che avverrà per l'appunto proprio qui in Senato: domani mattina, nella sala Zuccari alle ore 10,30, il Presidente del Senato - e a nome e per conto del Partito radicale non violento, transnazionale e transpartito rinnovo i ringraziamenti per questa sua disponibilità - inaugurerà un convegno che parlerà proprio di giustizia, non solo con i massimi

diciamo che non è proprio il miglior modo di aprire questa quarantott'ore, che inizierà domani mattina, di riflessione sullo stato della giustizia in Italia che - ripeto - ancora una volta la Corte europea dei diritti umani considera essere delinquente (non più abituale perché, protraendosi nel tempo, si potrebbe definire professionale). Il provvedimento licenziato dalla Camera

in questione. Molto spesso si dice che la toppa sia ancora peggio del buco. Questa è la conferma che, ancora una volta in corso d'opera, si insiste nel voler rattoppare un qualcosa che è radicalmente sbrindellato dalle stesse istituzioni che, a fasi alterne, sono riempite da questa o dall'altra parte politica. Le parti del codice penale che invece affrontano la questione a nostro avviso andrebbero affrontate in modo diverso. Abbiamo così cercato di elaborare,

e delle misure previste dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, cosiddetta «legge Gozzini». Tale argomento dimostra quindi al contrario come la legittimità della pena perpetua sia subordinata al fatto che non sia poi in realtà tale, che sia cioè limitata ed interrotta da benefici che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione dei valori condivisi dalla società e dall'ordinamento giuridico di riferimento; secondo l'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio secondo l'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d.: «ordinamento penitenziario») sono però previsti del reati, altrimenti cosiddetti «ostativi», per i quali si determina la possibilità di concedere i benefici previsti dalla «legge Gozzini» solo nei casi in cui i detenuti e internati per tali reati «collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*»; il che determina che la pena, per coloro che sono condannati all'ergastolo per uno o più dei suddetti reati «ostativi», è privata di ogni contenuto premiale orientato alla tensione rieducativa del condannato prevista dalla Costituzione, risultando di fatto una pena perpetua a scanso di una collaborazione con la giustizia (la qual cosa

poterla in qualche modo sanzionare a norma di legge, perché non abbiamo aggiornato il nostro ordinamento a buona parte di quelli degli Stati con i quali abbiamo fondato l'Unione europea o con cui facciamo parte nelle maggiori organizzazioni internazionali.

Ci sono altre sentenze della Corte costituzionale che - come già detto - abbiamo incluso nella fase premissiva di questo ordine del giorno, che lasciano tuttavia sussistere l'illegittimità dell'ergastolo in relazione all'aleatorietà, alla casualità e all'assoluta assenza di certezza che caratterizzano le ipotesi di concessione all'ergastolano dei benefici previsti dalla legge Gozzini, nonché della liberazione condizionale. La concessione di tali benefici è subordinata a circostanze fattuali mutevoli, non certe e non garantite; da apprezzamenti di fatto e prognosi di pericolosità fondati su valutazioni rimesse prevalentemente all'esame non del giudice ma di esperti, come tali esterni a quella «cultura della giurisdizione» le cui caratteristiche garantiscono la terzietà, la legalità, la giurisdizionalità della decisione in materia *de libertate*. Tali profili evidenziano quindi la contrarietà dell'ergastolo ai principi di stretta legalità e certezza della pena, nonché di giurisdizionalità necessaria di ogni misura restrittiva della libertà personale. Inoltre, il carattere fisso ed immodificabile della comminatoria edittale dell'ergastolo viola palesemente i principi di eguaglianza e ragionevolezza, di proporzionalità tra reato e pena, di individualizzazione della sanzione criminale, nonché di colpevolezza per il fatto. L'assenza, nel caso della comminatoria dell'ergastolo, di una cornice edittale entro cui modulare la risposta sanzionatoria adeguata al caso concreto, impedisce di fatto al giudice di esercitare la doverosa funzione di commisurazione della pena, in relazione alle caratteristiche del fatto di reato, del suo disvalore penale, dell'elemento soggettivo e degli altri criteri di cui all'articolo 133 del codice penale. L'ordine del giorno G100 si conclude con un impegno richiesto al Governo di rivedere le clausole di ostatività ai benefici premiali per i detenuti, in special modo dinanzi a condanne all'ergastolo, previste dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario citato poco fa, nella direzione di una loro armonizzazione con quanto previsto dalla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene, che quindi ci farebbe in qualche modo andare nella direzione dell'altro ordine del giorno fatto proprio dal Governo, e comunque a rivedere la pena dell'ergastolo nella direzione della sua abolizione. Tra l'altro, un dibattito del genere credo che possa essere arricchito da quanto potrebbe avvenire nelle prossime ore in Norvegia, dove abbiamo assistito ad una vera e propria strage e dove par di capire che la pena per quel tipo di reato sarebbe stata "limitata" a 21 anni di detenzione: probabilmente , una detenzione degna tanto quanto certa, ma che oggi pare i giornali ci dicano non essere ritenuta appropriata dalle autorità norvegesi. Si cerca quindi il modo di imputare di crimini contro l'umanità quell'atto avvenuto la settimana scorsa. Ciò deve essere seguito da vicino, perché sicuramente quanto avviene in quel Paese, che ha un tasso di democrazia probabilmente non così inficiato come quello è qualcosa dal quale trarre ulteriori spunti di riflessione sotto tutti i punti di vista, buoni ultimi anche l'amministrazione della giustizia e il sistema penitenziario. Concludo con un'ulteriore ripetizione di quello che, senza interruzione, come radicali proponiamo ormai da molti anni. Se il problema o i problemi della giustizia italiana, comunque siano - faccio notare che è stata proposta una riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario, salvo poi infilarla in un qualche cassetto della Commissione giustizia della Camera - devono comunque essere i problemi a cui va incontro il Presidente del Consiglio dei ministri, c'è un modo per cancellare qualsiasi tipo di problema. Inizia per l'appunto con la prima lettera dell'alfabeto ed è: amnistia. Amnistia e indulto sono l'unica risposta seria ai problemi della giustizia del nostro Paese, di 11 milioni di persone che, a vario titolo, sono coinvolte in questi processi. Di lì si può ripartire con una riforma radicale del nostro ordinamento giudiziario, che faccia gli interessi dei cittadini, quindi del diritto costituzionalmente codificato e di tutte le norme internazionali che l'Italia ha deciso di includere nei propri ordinamenti. Quello è il primo passo, ormai necessario, per liberarci anche dai gravami di tipo politico o politicante o politicista, che non aiutano la ricerca di una giustizia giusta per tutti.

quella che stiamo facendo, e prima di passare, domani, all'esame degli emendamenti, richiamo a me stesso

nel nostro Paese non può non essere richiamata nel dibattito e non può non influenzare le scelte, anche quelle di dettaglio, che noi compiamo con questa normativa, con questo disegno di legge. Siamo in presenza di un settore della pubblica amministrazione che va quotidianamente perdendo fette di credibilità. Sono tanti i cittadini che rinunciano, ce lo dicono le statistiche, ad incrociare il sistema giudiziario per ottenere giustizia e l'affermazione l'affermazione dei propri diritti. L'Unione europea con una certa frequenza ci censura, sia perché i processi sono lunghi e non arrivano nei tempi giusti perché le pene sono in qualche maniera incerte. Anche l'economia ne risente. I misuratori economici indicano che il settore pesa ed è forma di rallentamento

alle prese con dettagli, con questioni particolari - noi dell'opposizione le abbiamo definite, come noi le vediamo, come un dispiegamento di forze e di energie tese a tutelare l'impunità del *leader* della maggioranza - e tuttora comunque in attività

aggiornare i riti, eliminare i formalismi, rivedere sistematicamente la materia, sostenere il settore anche finanziariamente, considerato

ma quel che è ancora più grave è che, mentre questo processo così deprecabile e anche così improduttivo stava in piedi, non siamo stati capaci di avviare una riforma radicale, organica del sistema, o meglio ancora - lo devo dire - la maggioranza ha inteso, assumendosene una responsabilità

E tuttavia, anche in questo contesto, che dovrebbe suggerire non più norme particolari ma tanta fatica concentrata sulla revisione del sistema, dispiace - e i colleghi lo hanno detto chiaramente

che l'uso di procedimenti che hanno relazione con i procedimenti in corso e per i quali si è arrivati ad una ad una sentenza definitiva costituisca un elemento che argina il tempo fisiologico entro il quale il dibattimento si deve svolgere, così come non mi sembra che l'acquisizione delle prove, attraverso questa modalità

quella modalità di acquisizione delle prove e la quantità di eventuali testimoni abbiano fatto venir meno anche una

che il processo potesse essere pianificato, pur in presenza di tanti possibili cavilli e di elementi di dilazione che permangono nella nostra normativa.

dei procedimenti per via delle prescrizioni. Voglio ripetere - perché ne sono profondamente convinto - che questo è il destino peggiore che possa avere un processo, avere un processo, che può concludersi con un elemento di soddisfazione maggior o minore per le parti: il non concluderlo proprio è davvero la sconfitta della giustizia. Noi siamo in una percentuale che purtroppo è assolutamente alta. Quindi,

Allunghiamo ed aggraviamo l'agonia della giustizia, incrociamo sempre più spesso i termini di prescrizione. Non facciamo un buon servizio. riassumo il mio intervento dicendo che al malato-giustizia questa normativa non offre non offre una abbreviazione dei tempi di guarigione, ma anzi li allunga, disegnando la cronicità della sua condizione.

Non si accorgono che, così facendo, i criteri di valutazione dell'ammissione delle prove sono diventati quattro. Perché? penale che viene modificato fa riferimento all'ammissione di prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. Questa è la prima categoria. Quindi la griglia è la pertinenza.

autorizza la citazione, escludendo le testimonianze vietate dalla legge - su cui siamo d'accordo - e quelle manifestamente sovrabbondanti. Nel Nel caso in cui si azioni l'articolo 468, non esiste più il criterio della pertinenza, ma si va al criterio della sovrabbondanza. Se invece non si aziona l'articolo 468, ossia la richiesta dell'autorizzazione alla citazione, ma le liste vengono presentate, si applica l'articolo 495. L'articolo 495 è quello che precede: gli atti preliminari al dibattimento in cui si ammettono le prove. In quella fase, secondo la modifica, sono ammesse le prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti. Nel

il giudice può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue, e voi aggiungete: «e manifestamente non pertinenti». Quindi la griglia a questo punto diventa duplice. Poi, improvvisamente, la griglia viene del tutto eliminata. Cioè,

il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove "che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte". Ossia, se sono richieste a prova contraria se sono richieste a prova contraria di prove già assunte non c'è nessuna griglia, né di pertinenza, né di superfluità. Niente. Devono essere ammesse.

intervengo per sollevare un problema in quest'Aula che ha gettato nell'angoscia e nel panico molte migliaia di famiglie in questi giorni, che stanno ricevendo una lettera delle finanze nella quale viene loro richiesto di restituire il «*bonus* bebè» ricevuto nel 2005 (un *bonus* di 1.000 euro). Questa è una seconda lettera

per annunciare loro che avevano vinto la lotteria di un *bonus* di 1.000 euro. Bastava che uno dei genitori si recasse all'ufficio postale più vicino per incassarlo. In un materiale allegato si stabiliva poi un tetto di reddito di 50.000 euro senza specificare però, come apprendiamo oggi, se si trattasse di reddito netto o lordo. Sarebbe bastata - si diceva - una semplice autocertificazione. Questo comprensibilmente ha creato caos, confusione e, probabilmente, ha indotto in errore alcune famiglie. Ora giunge questa seconda lettera di tutt'altro tenore (ed è anche questo che vogliamo denunciarlo), una lettera minacciosa che arriva dal Ministero del tesoro ed intima alle famiglie che non ne avrebbero avuto diritto, secondo gli accertamenti, la restituzione del *bonus* entro 30 giorni con un aggravio di 3.000 euro di sanzione amministrativa e la minaccia di una denuncia penale. quindi per scontato che vi sia dolo, con famiglie perbene trattate come delinquenti; questo crea, come ho detto, allarme e preoccupazione in persone oneste, che sono cadute in buona fede nella trappola propagandistica, mi si consenta, del precedente Governo Berlusconi. Un vantaggio che pertanto diventa una beffa. ragione sono qui, signora Presidente, a chiedere che il Governo venga in questa Aula a chiarire, riferendo cosa intende fare per sanare questa situazione davvero incresciosa che colpisce famiglie oneste e bisognose - spesso per una differenza di poche decine o centinaia di euro rispetto al tetto previsto

Le sarei grato se entro la seduta antimeridiana di domani, ultima operativa della settimana, fosse reso disponibile ai senatori il testo del nostro bilancio prossimamente in discussione, senza doverlo pietire di qua o di là. Ne va della nostra possibilità di intervenire in Aula con cognizione di causa. Senatore Molinari, certamente la Presidenza farà presente tale esigenza agli Uffici. Ricordo solamente che, come forse lei sa, martedì c'è stato un altro Consiglio di Presidenza per apportare alcune modifiche necessarie